Ricordo che i tempi del dibattito sono stati ripartiti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e comunicati all'Assemblea nella seduta antimeridiana.

più qualificata a dare informazioni su aiuti che non possono mancare in proporzioni adeguate alla gravità della situazione.

Signor Presidente, signori senatori, ringrazio il Senato della Repubblica per avere offerto l'opportunità di un confronto, che sarà certamente utile, aperto e costruttivo. Sono persuaso che la previsione di legge che impone al Governo di informare il Parlamento circa lo svolgimento delle missioni all'estero non debba essere interpretata come una mera *routine*, ma possa e debba costituire occasione per un confronto tra Governo e Parlamento sui temi della politica estera. Tale scambio è vitale per individuare l'interesse del Paese e cercare di promuovere quel consenso largo intorno alle scelte fondamentali della politica estera che costituisce una delle condizioni di forza e di vitalità dei sistemi democratici bipolari.

non gli aspetti di carattere militare, sui quali riferirà in Commissione difesa il Ministro della difesa, ma gli aspetti relativi allo scenario politico delle missioni internazionali voi mi consentirete anche di allargare il mio ragionamento ai principali temi della politica internazionale, con particolare riguardo, ovviamente, agli sviluppi e alle iniziative più recenti che hanno toccato il nostro Paese. Partirò proprio da un riferimento che mi sembra essenziale e che non ha nulla a che vedere con le missioni di carattere militare, cioè il Consiglio europeo che si è svolto il 21 e il 22 giugno scorso, che ha segnato un punto di svolta importante della vicenda continentale e il momento in cui si è posto fine a due anni di paralisi e di incertezza sulle sorti del processo di riforma dell'Unione Europea. Non avremo il Trattato costituzionale, ma avremo in breve tempo una riforma dei Trattati, una riforma che, credo, debba essere considerata seria, nelle condizioni e date, perché includerà le principali innovazioni relative al funzionamento delle istituzioni europee, che erano già previste nel testo del 2004. Il Consiglio europeo ha approvato un mandato chiaro e molto dettagliato per la Conferenza intergovernativa.

in modo preciso e corretto, la traduzione in termini giuridici del mandato deciso dal Consiglio europeo. Anche per questo è ovviamente nostro auspicio, oltre che intenzione, che non si tratti di una classica Conferenza intergovernativa dall'esito aperto e che preveda un vero e proprio negoziato: il negoziato si è già svolto ed è quello che ha condotto al difficile compromesso mediato da Angela Merkel al Consiglio europeo del giugno scorso. La Conferenza intergovernativa dovrà avere un carattere eminentemente tecnico e dovrà limitarsi a tradurre in un articolato compiuto le indicazioni del mandato. È convinzione del Governo italiano, così come della Presidenza portoghese, che non esistano spazi per riaprire i punti già concordati nel Consiglio europeo; intendiamo difendere l'insieme del mandato approvato, combattendo rischi di arretramento: questo è il principale obiettivo che l'Italia si propone nella Conferenza intergovernativa. Ciò consentirà - ed è questo il secondo obiettivo - tempi rapidi. Il nuovo Trattato di riforma dovrà essere firmato, in ogni caso, entro la fine del 2007, in modo da poter dedicare un anno intero alle ratifiche, prima della scadenza elettorale del 2009, perché i cittadini europei siano chiamati a votare nel quadro di istituzioni rinnovate più efficaci, più democratiche e più forti. Come tutti i compromessi, anche quello raggiunto dal Consiglio europeo ha avuto dei costi. D'altro canto, la storia dell'integrazione europea è storia di compromessi, di accordi, di passi graduali. Per chi avrebbe voluto, come l'Italia, maggiori progressi sulla via dell'integrazione politica, il prezzo pagato è stato (per riprendere le parole del Presidente della Repubblica pronunciate recentemente a Lisbona), la riduzione delle ambizioni costituzionali dell'Unione. Non è un prezzo di poco conto, e ne sono prova la rinuncia al termine "Costituzione" e ai simboli dell'Unione, insieme a vari punti di arretramento. Se la delusione è comprensibile negli ambienti, nei Paesi e tra le forze più impegnati nel senso dell'integrazione politica dell'Europa, tuttavia la valutazione d'insieme deve, a mio giudizio, essere positiva e ciò per due ragioni. La prima è una ragione essenzialmente politica: la paralisi europea è finita. Paesi chiave, anzitutto la Francia, dopo le elezioni presidenziali con Sarkozy alla guida del Paese, sono tornati nel gioco europeo con una funzione attiva. La seconda ragione è che il compromesso raggiunto preserva, comunque, la parte qualificante di quello che potremmo definire il legato costituzionale del 2004. Ciò è anche risultato di una battaglia coerente, condotta dal Governo italiano insieme ai Paesi che, in modo più attivo, si sono impegnati a favore della innovazione costituzionale: fra questi, la Spagna, il Belgio, l'Austria e numerosi Paesi europei. Le innovazioni istituzionali sono state largamente preservate: un Presidente del Consiglio europeo stabile, eletto per due anni e mezzo; un Alto rappresentante per gli affari esteri e la sicurezza, che ha perduto il nome di Ministro degli esteri europeo (che, a mio giudizio, sarebbe stato migliore) e tuttavia ha mantenuto le prerogative e le funzioni previste dal Trattato costituzionale: disporrà del Servizio delle relazioni esterne e sarà, al tempo stesso, Segretario del Consiglio e Vice presidente della Commissione. Dunque, una posizione assai rafforzata, che rappresenta, in modo felice, una sintesi tra la dimensione intergovernativa e quella comunitaria, che sono le due grandi dimensioni dell'integrazione politica dell'Europa. La Commissione esce politicamente rafforzata dalla riduzione del numero dei commissari e dall'elezione parlamentare del suo Presidente che, dunque, avrà una legittimazione simile a quella di un Capo di Governo nella dimensione continentale. A questo si aggiunge che il sistema di voto a doppia maggioranza, anche con quello slittamento temporale che alla fine ha consentito di superare il veto polacco, rafforzerà la capacità di decisione dell'Unione. L'estensione significativa del voto a maggioranza qualificata e delle procedure di codecisione sono anch'essi momenti di rafforzamento della capacità democratica di decidere dell'Unione; in particolare, il ricorso alla maggioranza qualificata in molte nuove politiche che hanno un valore fondamentale, come quella dell'immigrazione. Bisogna aggiungere la personalità giuridica dell'Unione, il mantenimento del carattere vincolante dei diritti, sebbene sulla base di una norma di rinvio e con una clausola *opt-out* per il Regno Unito, e le nuove disposizioni, a mio giudizio di grande rilievo, sulla solidarietà energetica, sul mutamento climatico, sulla difesa e sulle cooperazioni rafforzate. Insomma, il quadro è - lo ripeto - un quadro nel quale le nuove regole appaiono in larga misura preservate e nelle condizioni di essere alla base di una rinnovata stagione di integrazione. È indubbio che la Germania abbia svolto, insieme alla Francia, un ruolo particolare nella ricerca di questo compromesso, naturalmente dovuto non soltanto al grande peso che la Germania esercita, ma anche al ruolo di Presidenza che in questa fase così delicata è stato svolto dal Governo tedesco. Ma è indubbio che anche i Paesi che di più si sono battuti per preservare il Trattato costituzionale - fra questi l'Italia hanno svolto un ruolo importante nel creare le condizioni di un compromesso avanzato e il Governo ha potuto svolgere un'azione coerente a sostegno della mediazione tedesca anche grazie a quella posizione favorevole all'integrazione europea che nel nostro Paese fortunatamente unisce la grande maggioranza delle forze politiche che si sono espresse nella ratifica del Trattato costituzionale e poi nel conferire al Governo il mandato di difendere, nella misura del possibile, le riforme che nel Trattato erano contenute. Sottolineo questo aspetto, l'esigenza di coesione nazionale nelle scelte europee, perché dobbiamo essere consapevoli della fase in cui siamo entrati, una fase segnata da un forte ritorno degli Stati nazionali, anche sul tavolo europeo. L'Europa allargata funzionerà sempre di più sulla base di stimoli e iniziative di coalizioni flessibili tra i Paesi che vorranno, ma insieme sapranno, costruire una cooperazione più stretta in settori specifici. In questo senso, le aree d'interesse prioritario per l'Italia sono, anche guardando a possibili cooperazioni rafforzate, il governo economico nell'area dell'euro, la sicurezza e l'immigrazione: sono punti di cui discutere e sono punti su cui costruire un progetto nazionale per l'Europa e insieme una capacità di alleanze per perseguirlo nel quadro delle istituzioni comuni. In giugno, abbiamo anche potuto registrare un consenso europeo sulla battaglia promossa dall'Italia, relativa alla moratoria delle esecuzioni e per l'abolizione della pena di morte. Esiste oggi un impegno condiviso per la presentazione di una risoluzione alla 62a Assemblea generale delle Nazioni Unite. Come Governo e come diplomazia siamo da mesi impegnati nella costruzione di alleanze internazionali e per la presentazione della risoluzione. Registriamo progressi importanti, che ho avuto modo di constatare anche nel mio recente viaggio in Africa. Diversi Paesi africani, innanzitutto il Sud Africa, saranno certamente tra i *co-sponsor* di questa iniziativa. Il sostegno europeo all'azione italiana sulla moratoria della pena di morte premia la costanza dell'azione delle organizzazioni della società civile, che da tempo si battono per questo obiettivo, ma anche dell'azione svolta dal Parlamento, dalla diplomazia italiana e dal Governo. È, anche questo, dunque, un risultato da ascrivere al fatto che il Paese è unito in questa battaglia di civiltà, dimostrando un'armonia di intenti e una comunanza di fini che purtroppo non è così frequente nel nostro Paese. Attualmente, in ambito Unione Europea si stanno definendo gli ultimi dettagli del testo della risoluzione, sulla base di quello che abbiamo proposto al Consiglio affari generali del 18 giugno scorso. Il vero e proprio banco di prova sarà l'Assemblea generale, che si aprirà a New York il 25 settembre e che proseguirà nei mesi successivi. La risoluzione sulla pena di morte, dal punto di vista procedurale, dovrebbe prevedibilmente essere presentata dai Paesi dell'Unione Europea e con un numero significativo di *co-sponsor* verso la fine del mese di ottobre. Fino a quel momento resteremo impegnati, insieme alle altre capitali europee, in un'azione di sensibilizzazione dei potenziali sostenitori della risoluzione così da raggiungere il più ampio numero di sostegni di Paesi appartenenti a tutti i gruppi regionali. L'azione dell'Unione Europea coinvolgerà già nel corrente mese di luglio anche le principali ONG attive contro la pena di morte, poiché si è convenuto sull'utilità di coinvolgere tutte le espressioni della società civile internazionale impegnate nella lotta alla pena di morte, sia a Bruxelles che a New York, dove, in occasione dell'apertura dell'Assemblea generale, promuoveremo un grande incontro dei Paesi e delle organizzazioni favorevoli a questa battaglia. L'azione dell'Italia sul fronte della moratoria è una testimonianza del ruolo attivo e della capacità propositiva del nostro Paese alle Nazioni Unite, un ruolo che è stato confermato e rafforzato dalla nostra elezione al Consiglio di sicurezza nell'ottobre scorso e lo è ancora di più a seguito della successiva elezione del nostro Paese nel Consiglio sui diritti umani. L'azione complessiva dell'Italia a New York, come del resto a Ginevra, per quanto riguarda i diritti umani, ha sempre tentato di valorizzare, per quanto possibile, il coordinamento europeo nella convinzione che una maggiore coesione e maggiori responsabilità dell'Europa nella gestione della sicurezza internazionale siano una delle condizioni per un multilateralismo efficace. Permettetemi un'ultima notazione su questo. Per quasi mezzo secolo l'Italia è stata un Paese consumatore di sicurezza prodotta e garantita da altri. Nella rigidità del mondo bipolare la nostra collocazione geopolitica rimediava anche alle nostre debolezze interne. Oggi, nel disordine post-bipolare, ciò non è più vero: dobbiamo produrre la nostra quota di sicurezza, assumendoci responsabilità nazionali dirette se vogliamo contribuire ad un sistema multilaterale che funzioni. Partecipare alle missioni internazionali, sulla base dei principi che riprenderò in conclusione, esprime il senso di questo cambiamento strutturale, e cioè quello di un Paese che intende partecipare, nei limiti delle sue possibilità, in modo attivo alla garanzia della sicurezza internazionale, da cui dipende anche la sicurezza del nostro Paese. Le dimensioni stesse della sicurezza, d'altra parte, si sono profondamente modificate rispetto al passato. Il vertice G8 di Heiligendamm è stato dominato da due nuove dimensioni della sicurezza: il rischio ambientale e i rischi legati agli squilibri economici globali, alle crescenti disuguaglianze, con particolare attenzione ai temi del sostegno allo sviluppo dell'Africa. Nella lotta al cambiamento climatico le posizioni di partenza divergevano notevolmente, in particolare tra gli europei e gli Stati Uniti. La mediazione della Presidenza tedesca ha tuttavia consentito qualche progresso: gli Stati Uniti sono passati da un sostanziale rifiuto del processo di Kyoto ad un attivo coinvolgimento nella ricerca di soluzioni che permettano di allargare gli impegni a Paesi come l'India e la Cina. L'accordo raggiunto al G8 riconosce alle Nazioni Unite il ruolo di principale foro negoziale. Le iniziative americane, tra cui una conferenza internazionale, dovranno portare a definire entro il 2008 un *global framework* per poi confluire in un accordo globale entro il 2009. Nell'avvio di questo processo peseranno le decisioni assunte dal Consiglio europeo le decisioni del Canada e del Giappone che, come è noto, impegnano a dimezzare le emissioni entro il 2050. In materia di sviluppo dell'Africa il G8 ha confermato e rafforzato gli impegni internazionali a favore degli Obiettivi del Millennio. È un terreno, quello dei livelli di aiuto pubblico allo sviluppo, su cui l'Italia si trova in chiara difficoltà per i tagli operati negli anni passati. Il Governo è riuscito a invertire la tendenza con la finanziaria del 2006 economico-finanziaria, intende consolidare la tendenza alla crescita nel 2007. A questo riguardo, mi sembra opportuno aprire una parentesi su un aspetto non secondario ed anzi qualificante del modo in cui il Governo interpreta il ruolo dell'Italia nel campo delle relazioni internazionali. Mi riferisco alla cooperazione allo sviluppo: gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 2007 hanno comportato un notevole incremento dei fondi ad essa dedicati, passati dai circa 380 milioni di euro del 2005 a oltre 600 milioni. A tale cifra devono poi aggiungersi i fondi destinati dal Governo all'azione di cooperazione in Afghanistan, Libano e Sud del Sudan, pari ad ulteriori 55 milioni di euro. Tale aumento ha rappresentato un segnale indubbio della rilevanza che il Governo intende attribuire all'attività di cooperazione. Si tratta, peraltro, di una chiara indicazione della determinazione a rispettare gli impegni assunti in sede ONU e Unione Europea, impegni che prevedono un costante aumento della percentuale di aiuto pubblico allo sviluppo sul PIL al fine di raggiungere l'obiettivo dello 0,7 per cento nel 2015. In questo senso sono chiare le previsioni del DPEF con uno stanziamento complessivo per la cooperazione che consentirà di raggiungere lo 0,33 per cento del PIL nel 2008, lo 0,42 l'anno successivo e lo 0,51 nel 2010. Si tratta di impegni molto rilevanti

rappresentano una condizione fondamentale per una crescita equilibrata, per una riduzione delle disuguaglianze ed anche per poter governare in modo efficace e giusto i grandi flussi migratori e i grandi problemi della sicurezza. Nell'immediato, attraverso l'aumento dei fondi stabilito dalla legge finanziaria in corso, è stato, tra l'altro, possibile riprendere il versamento dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali, che aveva raggiunto il livello minimo con notevole perdita d'immagine per il Paese, assicurare un rinnovato finanziamento alle organizzazioni non governative e mettere in opera una ripresa consistente degli aiuti bilaterali a gestione diretta. Non da ultimo, la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri è stata in grado di assolvere all'impegno di versare la quota prevista al Fondo globale contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e la malaria (quota che era arretrata rispetto a quanto era dovuto nel 2005), mentre il Governo si è impegnato ad erogare le successive somme promesse, consentendo all'Italia di riprendere con qualche credibilità la sua iniziativa a favore dei Paesi più svantaggiati. Per tornare al Vertice G8, proprio ad Heiligendamm è emerso un messaggio significativo in tema di lotta alle grandi endemie, confermando gli sforzi verso l'obiettivo dell'accesso universale alle cure per l'AIDS e il rifinanziamento del Fondo globale. Ai *partner* G8 il Presidente del Consiglio aveva già anticipato la volontà di riportare in linea, com'è poi avvenuto in occasione dell'assestamento di bilancio, il contributo italiano al Fondo globale. Il G8 si è, infine, impegnato a sostenere il rafforzamento delle istituzioni africane, inclusi gli organismi di sicurezza regionali e in questo ambito è stata approvata la proposta italiana di costituire una rete di centri di formazione di *peacekeeper* africani. L'importanza che l'Italia attribuisce agli sviluppi del continente africano è stata confermata dalle scelte bilaterali, tra cui la recente visita del Capo dello Stato in Ghana, la visita che ho compiuto insieme al ministro Bonino in Sudafrica, anche insieme ad un'importante missione imprenditoriale, seguita dalle tappe di lavoro in Mozambico e nel Congo. Il Governo ritiene che questa attività bilaterale sia funzionale alla preparazione del vertice Europa-Africa, che dovrà tenersi, dopo un'interruzione di ben sei anni, e che rappresenterà, credo, l'appuntamento più rilevante nel corso degli ultimi mesi dell'anno. È evidente che l'Europa è in un rischioso ritardo, specie se consideriamo l'attivismo della Cina e degli Stati Uniti, in un continente decisivo per la lotta alla povertà, per i problemi migratori e per le questioni emergenti. Il nuovo impegno di Parigi sulla questione del Darfur, appoggiato da Londra, ma anche da Roma, potrebbe segnare un salutare risveglio. Passo ora al principale evento internazionale promosso dall'Italia nelle ultime settimane, e cioè la Conferenza sulla *Rule of law* in Afghanistan, che si è svolta il 2 e il 3 di luglio. Come sapete, la Conferenza di Roma ha visto la partecipazione di 26 delegazioni di Paesi ed organizzazioni internazionali gli interventi del presidente afghano Karzai, del segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon, del Segretario generale della NATO, della Presidenza di turno dell'Unione Europea, di molte altre autorità di Governo, di rappresentanti di organizzazioni non governative, di organismi e di agenzie internazionali. Al di là del livello della partecipazione, che indica di per sé l'importanza attribuita dalla comunità internazionale alla riunione di Roma, ritengo importante sottolineare la concretezza dei risultati raggiunti. La Conferenza ha permesso di costruire un nuovo consenso da parte delle autorità afghane e della comunità internazionale su un punto chiave: la costruzione dello Stato di diritto come condizione della convivenza civile e politica in Afghanistan e come presupposto della stabilizzazione del Paese. Non si è trattato di un consenso retorico. Su questa base e sulla base dell'impegno afghano alla presentazione di un piano sulla giustizia, controllato e monitorato internazionalmente, sono stati raccolti nuovi finanziamenti per complessivi 360 milioni di dollari, un ammontare superiore alle aspettative, che è testimonianza - direi in questo caso concreta - del successo della Conferenza. Nello stesso tempo, la Conferenza è stata anche occasione per una discussione politica sulle prospettive della presenza internazionale in Afghanistan. È evidente che la vera battaglia da vincere per il Governo afghano e per la comunità internazionale è quella del consenso e della fiducia della popolazione afghana. È un punto centrale, su cui il Governo italiano richiama l'attenzione da mesi, in sede ONU e in sede NATO, con la credibilità che ci deriva dal fatto di figurare tra i Paesi maggiormente impegnati nella missione ISAF su mandato del Consiglio di sicurezza. Tuttavia, siamo convinti che questa insistenza debba continuare, dal momento che è evidente che, senza progressi concreti e rapidi nelle condizioni di vita degli afghani, non si riuscirà a garantire la stabilità del Paese. È altrettanto evidente quanto sia importante assicurare che le operazioni di contrasto al terrorismo, per quanto necessarie ai fini della sicurezza, non continuino sistematicamente a causare vittime tra la popolazione civile. Si tratta di danni e di vittime inaccettabili sul piano morale e che, nello stesso tempo, finiscono per compromettere la stessa immagine della presenza internazionale e per indebolire il Governo e le istituzioni democratiche dell'Afghanistan. Su questo tema, anche per iniziativa italiana, vi è stato un confronto nelle sedi internazionali, allo scopo di trovare un equilibrio migliore fra esigenze di sicurezza, di sicurezza, di ripresa civile del Paese, di difesa e di tutela delle popolazioni afghane. Sono temi di cui si è discusso anche nella Conferenza di Roma. Sono temi su cui il Governo italiano continuerà ad impegnarsi in sede internazionale, anche nella prospettiva di quella Conferenza per la pace in Afghanistan che rimane un nostro obiettivo strategico. Com'è noto, il Paese è impegnato anche su altri fronti. In alcuni casi il nostro impegno militare di sicurezza si colloca nel quadro di operazioni NATO su mandato delle Nazioni Unite, com'è il caso della nostra oramai decennale presenza nella KFOR in Kosovo, tema su cui tornerò dopo e che si presenta come uno dei punti più delicati nell'agenda attuale della politica internazionale. Più frequentemente, siamo impegnati nell'ambito di missioni di pace dell'ONU, come nel caso dell'UNIFIL, ma anche di altre missioni mediorientali (*United Nations Truce Supervision Organization*), della forza di *peacekeeping* a Cipro e della missione di monitoraggio alla frontiera tra India e Pakistan. Sempre più spesso, inoltre, partecipiamo a missioni promosse dall'Unione Europea, come in Bosnia, nel Sudan, nel Congo o in altre aree del Medio Oriente. Ho avuto modo in passato di illustrare il contenuto di tali missioni al Parlamento. Preferisco concentrarmi, dopo aver parlato dell'Afghanistan, sulla missione UNIFIL in Libano, visto il ruolo svolto dall'Italia, che ne ha il comando e che è stata senza alcun dubbio il principale Paese promotore di questa iniziativa internazionale. La missione internazionale in Libano è, in effetti, diventata uno dei banchi di prova fondamentali della possibile efficacia di un'azione internazionale in un quadrante decisivo come quello del Medio Oriente. A quasi un anno dal rafforzamento di UNIFIL, la significativa presenza internazionale del contingente ONU (oltre 13.000 militari) ha permesso alle legittime autorità libanesi, per la prima volta in trent'anni, di riprendere il controllo del territorio del Paese a sud del fiume Litani. Non va dimenticato che lo spiegamento di UNIFIL, rafforzata nell'estate del 2006, è stato essenziale per il cessate il fuoco, per la difesa della democrazia libanese e per consentire l'interruzione del conflitto che fu provocato da Hezbollah, ma che Israele ha gestito - come dimostrano i lavori della Commissione Winograd - compiendo notevoli errori. Analizzato un anno dopo e considerate le ricostruzioni della crisi del 2006, lo spiegamento del contingente internazionale è stato una decisione utile e giusta. Tuttavia, sarebbe perfettamente inutile nascondersi che la situazione sul terreno resta quanto mai complessa e a forte rischio. La tesi del Governo italiano è sempre stata che la missione internazionale non avrebbe potuto da sola risolvere i problemi del Paese in assenza di un processo politico interno e di un processo di distensione regionale. Vi sottopongo alcuni elementi di valutazione su questi due punti. Sul piano della sicurezza continuano a preoccupare le informazioni sul contrabbando di armi che affluirebbero in Libano dalla Siria, soprattutto - bisogna dirlo - al di fuori dell'area di responsabilità di UNIFIL, nonostante il divieto imposto dalla risoluzione 1701. La presentazione al Segretario generale, lo scorso 26 giugno, del rapporto redatto dalla missione LIBAT, che aveva il compito di verificare la situazione dei confini libanesi, fa stato di un livello di controllo dei confini tra Libano e Siria insufficiente a consentire un'efficace prevenzione. L'attacco del 24 giugno scorso contro un convoglio UNIFIL nel Sud del Libano, in cui hanno perso la vita sei caschi blu spagnoli e colombiani, ha confermato che il compito del contingente internazionale non è certo esente da rischi. Il Governo italiano ha predisposto misure di massima sicurezza per i nostri soldati. L'Italia è consapevole dei rischi, ma è anche conscia della validità dell'azione svolta dal nostro contingente nel Libano meridionale. Conferma tale validità la richiesta del Governo Siniora a fine giugno di estendere di un anno, fino al 31 agosto 2008, e senza emendamenti il mandato di UNIFIL. Ne discuteremo nel corso del mese di agosto nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Cresce intanto, dopo gli scontri ancora in corso nel campo profughi di Nahr el-Bared tra le forze armate libanesi e le milizie di Fatah al-Islam, il timore di un allargamento a macchia di leopardo dei focolai di tensione tra le forze armate libanesi e i movimenti di matrice estremista, in parte palestinesi, in parte provenienti da altri Paesi arabi, che hanno messo radici all'interno dei campi profughi palestinesi. La situazione interna libanese resta quindi assai critica. L'omicidio lo scorso 13 giugno del deputato della maggioranza Walid Eido fa temere una ripresa della stagione degli assassini politici dopo l'istituzione del tribunale internazionale per i responsabili dell'assassinio di Hariri. È decisivo, di fronte ai tentativi di destabilizzazione del Libano, rafforzare il sostegno della comunità internazionale al Governo Siniora, cercando di favorire il superamento di una paralisi politica interna in corso dal novembre scorso, ossia dalle dimissioni dall'Esecutivo Siniora dei cinque ministri di confessione sciita. Le aspettative di un accordo per la formazione di un Governo di unità nazionale quale via d'uscita dalla crisi in atto non si sono per ora concretizzate e potrebbero essere ulteriormente complicate dall'avvicinarsi della scadenza presidenziale. Il mandato dell'attuale Capo dello Stato giungerà a termine il 24 novembre prossimo e il primo scrutinio avrà luogo il 25 settembre. La ricerca di una figura di compromesso, che il patto non scritto del 1943 prevede sia ancora un cristiano maronita, appare ardua. La maggioranza di Siniora teme che concessioni alle forze dell'opposizione su tale terreno possano portare alla presidenza un'altra figura marcatamente filosiriana, mentre l'opposizione ha già dichiarato che, in mancanza di un accordo, non favorirà il raggiungimento del *quorum* per l'elezione del nuovo Capo dello Stato. È dunque evidente che la situazione appare complessa e che anche interferenze esterne continuano a costituire un forte ostacolo all'avvio di un positivo dialogo. Da questo punto di vista è stata positiva l'iniziativa assunta dalla Francia, anche se la Conferenza di La Celle Saint Cloud, promossa dal 14 al 16 luglio scorso, che pure ha rappresentato un passo importante, tuttavia non ha rappresentato un passo sostanziale. Si è trattato, per la prima volta dopo vari mesi, di un incontro a cui hanno partecipato i rappresentanti politici di tutti gli schieramenti libanesi, incluso Hezbollah, invitati dal Governo Sarkozy. Ma la mancata intesa sul documento politico conclusivo non è stata certo un segnale incoraggiante. Il Governo di Parigi intende tuttavia continuare in questo impegno, anche con una visita del Ministro degli esteri francese a Beirut. Si tratta di un impegno positivo al quale l'Italia è pronta a dare anche il suo contributo. In questo quadro, che è certamente rischioso, sembra emergere almeno una comune consapevolezza, che la soluzione dell'attuale crisi del Libano continua ad essere condizionata da decisioni che vengono prese al di fuori del Libano, in modo particolare in Iran, per la forte influenza che esso esercita su Hezbollah, ma anche in Siria, dato che quel Paese non sembra avere rinunciato alle pretese di influenza sul Libano, e in Arabia Saudita per i forti legami con il Libano e con la famiglia Hariri e per la difesa che l'Arabia Saudita esercita degli interessi sunniti in Libano. Anche in questo senso è in corso una iniziativa della diplomazia europea. Sia la Francia che la Spagna che la Germania si stanno adoperando attraverso missioni politiche e diplomatiche per esercitare una pressione sui Paesi interessati allo scopo di favorire un'intesa. Resta cruciale in questo quadro l'atteggiamento siriano; non è chiaro quale sistema di incentivi e di disincentivi potrebbe spingere la Siria ad associarsi in modo cooperativo ad uno sforzo di stabilità del Libano, ma è fondamentale continuare a spingere Damasco in questa direzione ed è un impegno al quale non può sottrarsi nessun Paese che voglia lavorare per la stabilità in quella parte del mondo. L'instabilità del Libano si connette all'acutizzarsi della crisi palestinese dopo il violento scontro tra Hamas e Fatah a Gaza. Lasciatemi dedicare alcune riflessioni a questo tema che continuerà ad assorbire le energie dell'Italia, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e dei Paesi arabi. La presa violenta del potere a Gaza da parte di Hamas, nel giugno scorso, ha posto fine alla fragile esperienza del Governo di unità nazionale palestinese, nato dagli accordi della Mecca e appoggiato dal Quartetto. La guerra civile intrapalestinese ha segnato una drammatica separazione tra Gaza e la Cisgiordania, con le implicazioni umanitarie che sono sotto gli occhi di tutti. Il 18 giugno il Consiglio dei ministri degli esteri dell'Unione Europea ha espresso forte preoccupazione per questi sviluppi e una ferma condanna per il colpo di mano militare di Hamas. Siamo oggi di fronte ad una spaccatura sia politica che territoriale della popolazione palestinese, con tutti i rischi che ciò comporta per la prospettiva di uno Stato democratico funzionante e unitario. È evidente che una futura ricomposizione sarà indispensabile per poter salvaguardare la prospettiva di una pacificazione fondata su due Stati indipendenti. La gravità della crisi ha d'altro canto condotto ad una ripresa di attivismo diplomatico, con alcune opportunità che dovranno essere colte rapidamente e gestite con lungimiranza. Anzitutto, la formazione del Governo guidato da Salam Fayad ha incoraggiato il dialogo bilaterale tra il premier israeliano Olmert e il presidente Abbas. Israele ritiene di poter finalmente contare su un interlocutore palestinese affidabile. Si sono avuti alcuni primi risultati concreti: l'accelerazione del rilascio dei 250 prigionieri palestinesi, di cui erano stati già concordati i nomi; l'alleggerimento della pressione dei posti di blocco in Cisgiordania; la ripresa parziale di trasferimenti finanziari e la sospensione dei mandati di cattura contro 178 esponenti di Fatah. Erano richieste attese da tempo, ma hanno anche segnato una svolta nel rapporto bilaterale. Per poter consolidare questa svolta dovranno tuttavia seguire, come ha auspicato il presidente Prodi nel corso della sua recente visita in Israele e nei territori, altre concessioni concrete, in particolare sulla libera circolazione delle persone, che permettano di alleviare la condizione della popolazione palestinese, rafforzandone la *leadership*. In secondo luogo, e come ha confermato il vertice a quattro di Sharm el Sheikh di fine giugno, a cui hanno partecipato Mubarak, il Re di Giordania, il primo ministro Olmert e il presidente Abbas, Egitto e Arabia Saudita hanno deciso di impegnarsi direttamente e più attivamente per sostenere la ripresa del dialogo bilaterale tra Israele e il nuovo Esecutivo palestinese. La gravità della crisi di Gaza ha insomma consolidato gli spazi di convergenza tra Israele e una parte delle forze palestinesi, i principali attori regionali che avevano in questi mesi sostenuto il rilancio dell'iniziativa di pace della Lega araba. Si è inserito in questo quadro, infine, il discorso pronunciato il 16 luglio dal presidente Bush che ha in particolare avanzato la proposta di convocare in autunno una conferenza internazionale, a cui parteciperebbero le parti, i Paesi vicini, gli Stati Uniti e i rappresentanti dei Paesi che sostengono la soluzione dei due Stati. Come sapete, la necessità di una Conferenza internazionale per il rilancio del processo di pace figura da tempo tra le priorità diplomatiche indicate dall'Italia e dall'Europa. È una delle proposte avanzate nella lettera aperta dei dieci Ministri degli esteri europei, dell'Europa mediterranea e meridionale, tra cui la Francia, la Spagna e l'Italia, e rivolta al nuovo inviato del Quartetto, Tony Blair. Ed è una proposta rilanciata nella risoluzione sul Medio Oriente, approvata a larghissima maggioranza dal Parlamento europeo il 12 luglio scorso che, fra l'altro,

riprende la lettera dei dieci ministri a Blair, definendola un messaggio incoraggiante, di sostegno alla sua missione, oltre che diversi concetti contenuti nella lettera. Ma si vede che quello è un ambiente lontano, dove la discussione è forse più serena. Chi lo sa! Comunque, è sempre possibile cambiare idea. Lo stesso presidente Prodi ed io abbiamo ribadito a Tony Blair, negli incontri a Roma della settimana scorsa, il pieno appoggio dell'Italia: l'incarico del Quartetto all'ex Primo Ministro britannico che dovrà, in particolare, promuovere il rafforzamento della struttura statale Dell'Autorità palestinese, segna di per sé un aumento del profilo europeo nella gestione della crisi mediorientale. Nella proposta americana, la Conferenza internazionale avrà l'obiettivo di sostenere il processo bilaterale in corso, nella prospettiva della formazione di uno Stato palestinese, che sia accettabile anche per Israele ed abbia continuità territoriale. Le questioni più delicate sullo *status* finale verrebbero rinviate ad un momento successivo. Formato e ambizioni della Conferenza verranno discussi e chiariti nel corso delle prossime settimane. Il Governo italiano ha commentato con favore questo impegno americano a favore di un accordo di pace israelo-palestinese. Nel frattempo, la proposta di una Conferenza internazionale è stata accolta in termini positivi, anche se con molte cautele da Israele, dalla Lega araba e dall'Arabia Saudita. Un appoggio esplicito alla proposta di Bush è stato espresso dal Quartetto (il che vuol dire quindi, oltre che dagli Stati Uniti e dall'Europa, anche dall'ONU e dalla Russia) con la dichiarazione del 19 luglio scorso, dove si sostiene che la Conferenza dovrà fornire un sostegno diplomatico a negoziati bilaterali, che permettano di progredire con successo verso la creazione di uno Stato palestinese. Il Quartetto ha anche auspicato un ampio coinvolgimento dei Paesi della regione, ribadendo l'importanza dell'iniziativa di pace della Lega araba. L'Italia si impegnerà in tal senso, in particolare per favorire una partecipazione dei Paesi arabi, inclusi quelli che non hanno relazioni diplomatiche con Israele: in particolare, l'Arabia Saudita. La mia analisi è che esista una effettiva opportunità di avvicinamento tra Israele ed i Paesi arabi cosiddetti moderati, ma potrà essere colta solo se effettivamente si faranno progressi sul cammino della pace per i palestinesi e gli israeliani. Più in generale, dunque, la nostra azione diplomatica su questo tema cruciale si muove su tre pilastri fondamentali: anzitutto, il sostegno al presidente Abu Mazen, agli sforzi per dare vita ad un Governo di unità nazionale prima ed oggi, dopo la crisi di Gaza, al Governo presieduto da Salam Fayad. Ho visto che nelle polemiche condotte la generosità in questi giorni si è messo in dubbio il sostegno dell'Italia, in particolare del Ministro degli affari esteri, al Presidente palestinese. Ora, io penso che questo sarà un argomento che farà sorridere i palestinesi, nel senso che tutti sanno (almeno loro) quanto sia forte il legame, non solo politico, ma anche - consentitemi questa digressione - personale. Io fui inviato nei territori palestinesi dall'Organizzazione internazionale socialista allo scopo di incoraggiare il presidente Arafat a nominare Abu Mazen primo ministro ministro e svolsi la mia missione nel segno non soltanto di un costante impegno politico nella Regione - che a vario titolo mi impegna da molti anni - ma anche nel segno di una forte solidarietà personale verso uno degli esponenti che, senza dubbio, ha dato il contributo più coraggioso alla prospettiva della pace. Forse Forse lo si sarebbe potuto sostenere con maggiore generosità quando egli era al Governo, prima che si svolgessero le elezioni, che furono poi vinte da Hamas, forse anche perché allora non era stato sostenuto con sufficiente generosità dalla comunità internazionale. Chiudo questa digressione di carattere personale, che poi è una testimonianza. Sostenere Abu Mazen significa intensificare ed accelerare gli aiuti ed anche incoraggiare le riforme fondamentali per quanto riguarda lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione. Sono parametri cruciali per rafforzare l'immagine e la legittimità della *leadership* palestinese presso i palestinesi e quindi per allargarne le basi di consenso. L'appoggio che noi forniamo al presidente Abbas si combina alla convinzione che sarà anche necessaria una ripresa del dialogo politico interno ai palestinesi, in uno spirito di ricomposizione nazionale che possa prevenire la spaccatura permanente, politica e geografica, tra Gaza e la Cisgiordania. È appunto questa la linea sostenuta dai Governi dell'Europa mediterranea, di destra e di sinistra, e dal Parlamento europeo, con voto quasi unanime. In secondo luogo, l'Italia ha sostenuto e sostiene che sia anche nell'interesse di Israele garantire alla parte palestinese risultati concreti, tangibili e immediati. Si sono registrate alcune prime decisioni positive ma dovranno seguirne altre, in particolare sulla mobilità delle persone e per quanto attiene al congelamento degli insediamenti, oltre che alla rimozione dei cosiddetti avamposti illegali, come si dice nell'ultima raccomandazione del Quartetto. Si tratta di passi essenziali per accrescere la fiducia tra le parti, per rafforzare la *leadership* palestinese e per riaprire quell'orizzonte politico in direzione di un futuro Stato palestinese senza il quale, inevitabilmente, le posizioni più estremistiche continueranno ad avere forza e consenso tra i palestinesi. Infine, è decisivo evitare una crisi umanitaria a Gaza.

I rapporti delle Nazioni Unite su Gaza indicano la realtà di un territorio vicino al collasso, dove l'esasperazione della gente rischia di raggiungere livelli incontrollabili. È uno scenario che prelude al rischio di un'ulteriore radicalizzazione, il che certamente sarebbe assai rischioso. A me sembra evidente che mentre sosteniamo con convinzione l'Esecutivo di Salam Fayad dobbiamo porci il problema di come evitare un'ulteriore radicalizzazione e una frattura infrapalestinese, che alla lunga non favorisce la pace, né garantisce la sicurezza di Israele. Era questo lo spirito di un passaggio della lettera aperta dei dieci Ministri degli esteri dell'Unione Europea, che vi leggo: «Non bisogna spingere Hamas verso un'*escalation* estremistica. Bisogna riaprire la frontiera tra Gaza e l'Egitto. Bisogna facilitare il transito fra Gaza e Israele. Bisogna incoraggiare l'Arabia Saudita e l'Egitto a ristabilire il dialogo tra Fatah e Hamas».

Come vedete, questa lettera non propone, né ho mai proposto che la comunità internazionale apra negoziati diretti con Hamas. Ciò che si sottolinea è la necessità di evitare l'isolamento di Gaza, l'isolamento di Gaza, il rafforzamento del radicalismo di Hamas, di spingerla fra le braccia di Al Qaeda, e la necessità di incoraggiare la ripresa di un processo palestinese di riconciliazione nazionale. Queste sono le posizioni - ripeto - sostenute dall'insieme dei Paesi europei del Mediterraneo e dal Parlamento europeo,

Siamo impegnati con i nostri *partner* europei e internazionali a mettere fine al conflitto israelo-palestinese; sosteniamo il dialogo tra le parti; siamo a favore di una Conferenza internazionale che faccia seriamente avanzare il processo negoziale verso due Stati. Auspichiamo, nello stesso tempo, che la logica dello scontro tra i palestinesi possa essere superata anche attraverso un dialogo che premi le posizioni favorevoli alla pace. L'alternativa, una guerra civile su vasta scala, sarebbe una tragedia per i palestinesi e anche una seria minaccia per la sicurezza di Israele. Israele. Mi sia consentito, da ultimo, parlare brevemente della situazione del Kosovo, l'altro tema di grande attualità che ci coinvolge direttamente per la presenza dell'Italia in quel Paese con 2.000 militari, con la responsabilità di una parte del Kosovo e per la nostra presenza nel Gruppo di contatto e nel Consiglio di Sicurezza. Si tratta quindi di una questione che ci coinvolge a vario titolo e che rappresenta un banco di prova assai complesso per la comunità internazionale. Come è noto, l'Italia ha espresso un sostegno alla proposta avanzata dal negoziatore delle Nazioni Unite, Martii Ahtisaari, che prevede una sorta di indipendenza sotto supervisione internazionale del Kosovo, da realizzarsi, in particolare, sotto la responsabilità dell'Unione Europea. Abbiamo lavorato sempre perché ad una soluzione di questo tipo si potesse e si possa arrivare attraverso la condivisione delle parti interessate, innanzitutto i serbi e i kosovari. Abbiamo lavorato essenzialmente per aiutare la Serbia, che è un Paese amico e a noi vicino, a chiudere l'ultimo capitolo di una vecchia e drammatica storia, in modo da concentrarsi su una nuova agenda, quella della sua piena integrazione in Europa. In questo senso l'Italia si è battuta perché riprendessero i negoziati tra Unione europea e Serbia per un accordo di associazione, ciò che finalmente è accaduto. Siamo giunti nelle scorse settimane a uno snodo decisivo. Nel Consiglio di Sicurezza non ci sono le condizioni per approvare una nuova risoluzione. La minaccia di un veto russo e la pressione che è venuta da altre parti per un'accelerazione unilaterale del processo hanno messo l'Europa in una situazione difficile. È importante che si sia riusciti intanto a raggiungere un accordo per evitare lo scontro alle Nazioni Unite Unite e lo scenario drammatico di un veto e per rilanciare un negoziato diretto tra le parti che dovrebbe avvenire sotto l'egida di una *trojka*:

se il rappresentante europeo dovesse essere un rappresentante dei quattro Paesi che fanno parte del Gruppo di contatto. L'Italia si è battuta perché il rappresentante europeo sia un rappresentante dell'Unione Europea Paese parte del Gruppo di contatto, questa posizione è stata apprezzata. Alla fine si è deciso

Noi speriamo in questo negoziato bilaterale, cui l'Europa dovrà dare un grande impulso, considerata la sua funzione chiave nella Regione. Il futuro della Serbia non può prescindere dall'Unione europea, né può esservi un'indipendenza del Kosovo senza l'assistenza europea: la chiave, dunque, è in Europa e l'Europa deve riuscire ad esercitare la sua autorevolezza, spingendo verso un accordo che ponga fine, in questo modo, al lungo conflitto balcanico. Ciò è essenziale per aprire non soltanto alla Serbia e al Kosovo, ma a tutti i Paesi dei Balcani occidentali la prospettiva di un'integrazione nell'Unione europea, l'unica prospettiva nella quale la lunga guerra civile balcanica potrà essere considerata conclusa. conclusa. Le missioni internazionali, quindi, sono parte della trama di una complessa politica estera che si misura con sfide difficili e cruciali cui l'Italia cerca di dare il suo contributo. Queste missioni sono coerenti con la scelta del nostro Paese, direi con il dettato costituzionale, con una Costituzione che impone al nostro Paese i vincoli che derivano dalla nostra adesione agli organismi internazionali. Queste missioni sono coerenti con la necessità di una forte assunzione di responsabilità, da cui dipende anche l'efficacia di una politica multilaterale che, se non produce pace e sicurezza, non serve a nulla.

nazionali, evidentemente connessi al mantenimento della pace nelle Regioni cruciali che interagiscono con il nostro Paese. Si tratta di criteri che devono trovare rispondenza nell'azione internazionale sul terreno, sul terreno, nonché di criteri che devono continuamente trovare conferma e sostegno nel Parlamento e nell'opinione pubblica.

nostri militari impegnati in missioni internazionali. Essi sono tra i più apprezzati in questo tipo di lavoro

militari siano apprezzati per il fatto che sanno combinare l'efficienza militare ad una grande capacità politica: creare la pace non è soltanto il compito di chi fa la sentinella contro i violenti, ma è anche il compito di chi sa disarmare gli animi e preparare le persone alla cultura della pace.

«Io spero che Rifondazione Comunista, il PDCI e i Verdi traggano il giusto insegnamento da quanto accaduto. Devono rendersi conto che il giochino di chi sta al Governo e poi va a fare i cortei per la strada non funziona più,

la realtà e a quella che è la discrasia all'interno della sua maggioranza per rilevare che, prima di chiedere e di auspicare l'unità

un Governo estremamente debole, che esprime tutta la sua debolezza in politica estera. Come possiamo noi condividere la politica estera da lei espressa quando, di fronte ad alcuni argomenti fondamentali, di fatto esistono questa discrasia e questa incapacità?

che è stato un rapporto speciale e che continua ad essere un rapporto speciale, dice veramente poco perché sostiene che, di fatto, è un fenomeno di ordinaria amministrazione. A me sembra, invece, che si debba affrontare e si debba dire con grande forza che il rapporto con gli Stati Uniti di America è un rapporto fondamentale, è un grande pilastro dell'Italia e dell'Europa. *(Applausi dal Gruppo FI)*. Non si può sottacere questo aspetto, che è fondamentale.

che ha pagato tante volte e che ha aiutato tanti popoli e oggi è nel mirino, signor Ministro, della Jihad globalizzata, il cui obiettivo - ecco perché riprenderò più avanti le considerazioni su Hamas ed Hezbollah

chiara da parte del Governo nei confronti dei rapporti transatlantici: non si può non considerarli un elemento fondamentale. Attraverso Hamas, Al Qaeda sta entrando nella Striscia di Gaza. Qui mi addentro veramente nel problema. Quando lei, signor Ministro,

a proteggere Al Qaeda e che attraverso i suo comportamenti sanguinari Hamas è diventata molto vicina ad Al Qaeda. Aggiunge, Abu Mazen: «Condanniamo le azioni di Hamas in quanto crimini contro il popolo palestinese. Non apriremo nessun dialogo»; invece lei, signor Ministro, in qualche modo, attraverso alcune affermazioni, riconosce o comunque dà una considerazione sia ad Hamas che ad Hezbollah. Quando dice che «sono forze che rappresentano il popolo», è chiaro che il

si deve essere in qualche modo coerenti rispetto ad una politica di avvicinamento nei confronti di questa posizione terroristica.

PIANETTA). Signor Ministro, tutte queste sono posizioni che indeboliscono la posizione dell'Europa e all'interno di questa la posizione dell'Italia. L'Europa non può indebolirsi, come non può rinunciare ai propri princìpi di libertà. L'Italia non può e non deve assumere posizioni equivoche nei confronti del terrorismo, perché il terrorismo è la negazione della dignità umana e i *kamikaze*

altro che avere dei rapporti preferenziali, dei rapporti storici: è questo che vogliamo? Abu Mazen dice che Hamas è connivente di Al Qaeda: «Hamas commette crimini sanguinosi contro il nostro popolo, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto». E' tutto ciò che vogliamo? Credo proprio di no! Credo proprio di no! L'Italia con queste posizioni del Ministro degli esteri accentua le proprie ambiguità.

non può non lasciare perplessi il fatto che la Farnesina non abbia né condannato la sanguinosa la sanguinosa posizione di Hamas a Gaza, né dato il suo appoggio al nuovo Governo costituito dal Presidente dell'Autorità palestinese; concludeva poi affermando nel flirtare con Stati *sponsor* del terrorismo occorre tener presente che oggi il nemico non sta solo al di là dei confini ma ce l'abbiamo anche noi in casa nostra.

estera sulla sicurezza di tutti i nostri concittadini ed è colpevole chi non considera questi atteggiamenti con responsabilità. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, in tema di politica estera il nostro Paese agisce da sempre rifacendosi ai dettami della nostra Costituzione, autorevole ed insuperabile nel rifiuto della guerra come mezzo di soluzione nelle controversie internazionali, in nome cioè di quelle disposizioni superiori che pongono l'Italia come soggetto attivo in sede internazionale e quale Paese di riferimento per lo sviluppo della pace. La presenza dei militari italiani al fianco di quelli di altri Paesi è sotto l'egida della Comunità internazionale; si rende doverosa, dunque, per due ordini fondamentali di motivi: in primo luogo, per rispettare gli accordi presi nell'ambito delle istituzioni europee e mondiali di cui l'Italia fa parte e nelle quali ha sempre avuto un ruolo preminente; luogo, per ragioni di ordine morale ed etico, in quanto milioni di persone - uomini, donne, bambini, vittime indifese - non possono essere lasciate in balia del proprio destino senza che che ci si adoperi in alcun modo per il ripristino di condizioni di normalità e affinché tutti quei popoli per anni oppressi da regimi autoritari possano valersi di istituzioni democratiche. Sono questi gli argomenti che rendono indispensabile la presenza dei nostri militari nelle zone in cui sono chiamati ad operare sulla base delle scelte di politica estera che oggi il ministro D'Alema ha inteso chiaramente ed efficacemente illustrare. L'Italia da sempre svolge, infatti, un ruolo di Nazione guida e, soprattutto negli accordi tra istituzioni mondiali, rappresenta un modello di responsabilità e di etica e un faro per tante vittime dell'oppressione. Il nostro ruolo e compito primario in politica estera deve essere quello di trasfondere a tutti i popoli oppressi da regimi autoritari la nostra idea di democrazia, il nostro senso di uguaglianza, la nostra voglia di libertà. Brevemente, colleghi, vorrei fare accenno al problema, oramai ultradecennale, del conflitto tra israeliani e palestinesi. La Conferenza di pace prevista in autunno potrebbe rivelarsi davvero un primo passo verso la soluzione dell'annosa questione mediorientale. È necessario, però, come afferma il Ministro della Farnesina, che in questa conferenza vi sia una rilevante cornice politica multilaterale e multinazionale che veda coinvolte tutte le massime potenze mondiali. È questa l'ottica sulla quale continuare a lavorare: quella delle scelte condivise e adottate in tavolo di concertazione e alla presenza delle parti in causa. non è mai stato, per tradizione, un Paese disinteressato alle questioni internazionali né tanto meno insensibile alle richieste di aiuto, da qualsiasi parte del mondo esse provengano. Non può, quindi, suscitare scandalo una politica di mediazione e di moderatezza in campo internazionale, come quella che guida l'azione di questo Governo. Mi avvio a conclusione e vorrei anticipare che il Gruppo dei Popolari-Udeur esprimerà sicuramente il voto favorevole alla mozione di maggioranza e intende così confermare il pieno appoggio alle linee di politica estera espresse dal Governo in materia di missioni internazionali. *(Applausi del

D'Alema ha detto cose importanti che condivido e vorrei segnalare alcune esigenze di maggiore dinamicità e di svolta su alcuni punti. Nello stesso tempo, non voglio sottrarmi a quello che ha detto il senatore Pianetta prima, quando ha accusato il ministro D'Alema di non aver parlato degli Stati Uniti che sono un pilastro della politica estera. Penso anch'io che gli Usa siano un pilastro della politica estera, tuttavia oggi dobbiamo fare i conti con il fallimento di questa politica estera e non

ha decretato il proprio fallimento nella zona più drammatica, importante e critica rispetto alle situazioni di difficoltà internazionali: il Medio Oriente,

rispecchia, quindi, il fallimento acclarato drammaticamente di fronte a noi di questa amministrazione; chiediamo agli americani di poter cambiare presto con una linea di cooperazione e di grande apprezzamento multilaterale, il contrario di quello che è stato in questi anni, il combattimento contro il terrorismo è diventato solamente una forma di guerra che ha alimentato nuova guerra. Questo è ciò che chiaramente noi oggi non possiamo più fare e che, in alcuni punti importanti della relazione del ministro D'Alema, viene fuori come esigenza per ricostruire e ridefinire nuove linee di pace.

stati ottenuti risultati positivi. Certo, si sono verificate situazioni difficili ed importanti con atti contingenti che dimostrano quanta è alta la tensione, ma che nello stesso tempo va governata e che i nostri soldati stanno governando bene insieme agli altri.

come ha detto giustamente il Ministro, con cui concordo ed anzi andrei più avanti, c'è bisogno di capire quali novità bisogna immettere, cioè il rapporto tra la necessità dell'unità politica

come lo è - questa è la nostra preoccupazione - non può che essere fonte di ulteriori minacce e di ulteriori tentazioni di vario tipo. Nelle tentazioni jihadiste possono cadere tanti giovani non solo palestinesi, ma anche altre forze e frange che possono essere tentate da questa soluzione. Il nostro obiettivo, perché UNIFIL continui a svolgere positivamente il proprio ruolo, è appunto favorire un complesso ambientale positivo, cioè l'unità politica di quel Paese, perché nessuna delle fazioni si faccia strumento di disegni altrui. E qui invito non

Che so, penso a quanto sarebbe importante che Israele, entro un complesso più ampio di discussione, restituisse le alture del Golan alla Siria: significherebbe che si è aperta un'altra era,

una fetta importante di palestinesi nella disperazione e nella volontà di creare ulteriori disperanti azioni che non porterebbero la pace (anzi, nemmeno Israele sarebbe più ulteriormente sicuro).

seria iniziativa politica, ossia la Conferenza internazionale. Bene: abbiamo aumentato le dotazioni ai nostri soldati (cui va tutto il nostro appoggio), ma prevale una realtà in cui la guerra è in un vicolo cieco; troppi troppi morti civili impediscono di creare - come si è detto - consenso e fiducia (anzi, si stanno sviluppando disperazione e grande rabbia contro l'Occidente). Il Ministro ha ripetuto spesse volte che la politica deve riconquistare il proprio ruolo: sono d'accordo. È stata quindi avanzata la proposta di dar luogo alla Conferenza internazionale; oggi, forse, dobbiamo compiere un atto in più: la soluzione diplomatica deve essere perseguita con forte determinazione, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, esterni e interni a quel Paese,

che sta rischiando di mettere in discussione la sicurezza dell'Europa. Questo è uno degli aspetti essenziali; certo, vogliamo fare i conti con la politica degli USA, ma quando si arriva allo scudo spaziale, essa rischia di rappresentare un ulteriore alimento alla tensione e - guarda caso - anche all'interno dell'Europa. L'Europa sarà forte e unita se saprà fare i conti con queste linee politiche.

Signor Presidente, abbiamo ascoltato una relazione del Ministro degli esteri che potremmo definire passionale; tuttavia, sappiamo che è una bugia, perché metà di questo emiciclo faceva fatica a rimanere lesto ad ascoltarla: non se per mancanza di contenuti o per il fatto che lo stesso Ministro ha difficoltà a proporre la politica estera di questo Governo.

con quel Gruppo che conosciamo, importante e determinante per il Governo, voce di quella sinistra estrema che ha preteso sempre la discontinuità. Nei rapporti internazionali vige la garanzia e l'affidabilità, ma uno Stato, secondo una parte della sua maggioranza, dovrebbe continuamente modificare i rapporti con la comunità internazionale. A noi ciò fa paura, per il semplice fatto che il suo Governo ha già dimostrato di essere "sindacato-dipendente".

che ci vedono presenti soltanto per portare un po' di giustizia e di civiltà: almeno, tali sono le determinazioni dell'ONU, della NATO e della Comunità Europea. Andiamo in Paesi dove

sulla giustizia, stiamo trasmettendo il nostro ordinamento giuridico e giudiziario, i nostri codici approdano in quel Paese. Impareranno a conoscere cosa sono le garanzie e cosa sono i diritti umani.

notare queste contraddizioni intrinseche della sinistra: a me risulta che, in ogni altro momento, la sinistra abbia sempre rivendicato la totale autonomia dei magistrati. In questo momento schiera addirittura il Capo dello Stato

Nonostante questo, la Lega non è mai stata legittimata, sempre da voi, perché noi vorremmo «sovvertire» l'ordine costituito. Soltanto perché a noi non sta bene questo Stato, così incapace di rispondere ai bisogni del Paese, uno Stato arcaico e dissipatore delle risorse - è sotto gli occhi di tutti - costoso e inefficiente. Noi vorremmo organizzarlo in modo più democratico e addirittura con autonomie diffuse, pensate un po', in una parola il federalismo. Questo però basta per non essere legittimati e non essere da voi riconosciuti. Ministro, partito riconosciuto e democraticamente eletto. A noi risulta che Hamas, oltre che essere un'organizzazione terroristica che si rifiuta di partecipare alla comunità internazionale perché non riconosce nemmeno lo Stato d'Israele, all'indomani della vittoria, abbia cacciato tutti i rivali del partito di Al Fatah: questa è democrazia? Hamas è inserita nella lista dell'Unione Europea che annovera tutte le organizzazioni terroristiche. Messa al bando dalla comunità internazionale, dovrebbe essere riconosciuta dal nostro Paese?

di questo, di affidabilità, di rischi e di terrorismo internazionale vorremmo ricordare un'altra cosa riguardo ad incresciosi episodi accaduti in questo Paese. Ogni tanto si va a mettere le mani su qualche Moschea e, guarda caso, succede quel che succede. Abbiamo capito, abbiamo visto a Perugia, anche in tal caso per indagini sommarie operate dai nostri magistrati, che non si insegnava l'integrazione o la cultura della pace, ma - a detta dei nostri magistrati e dei nostri inquirenti - si organizzava una scuola paramilitare. Si insegnava a pilotare dei *jumbo* - e immagino che si insegnasse solo a decollare perché probabilmente l'atterraggio non sarebbe neanche servito

assicurare alla giustizia i docenti, ma non ci preoccupiamo del Paese. E gli allievi che frequentavano quei corsi, come li dobbiamo considerare? In questo Paese cosa ci stanno a fare? Con che spirito vivono? Con lo spirito di integrazione? Abbiamo qualche dubbio. Trattiamo anche con questi, magari? O li rispediamo a casa, tutti, una volta e per sempre? Egregio Ministro, so per che per voi questo sarebbe un grave e difficile dilemma, ma le assicuro che la gente comune saprebbe subito cosa fare. Purtroppo, anche in relazione alla segnalazione che ci era stata fatta all'inizio della seduta dal senatore Mantovano, devo informare il Senato la situazione nel Comune di Peschici si è ulteriormente aggravata; ci sono quattro vittime, cinquecento persone vengono evacuate dalla Capitaneria del porto di Vieste per ora la situazione non sembra destinata a migliorare. Vorrei esprimere, a nome del Senato, il cordoglio di tutti noi alle famiglie degli scomparsi e la solidarietà alle vittime di questa tragedia, dovuta allo spaventoso incendio che ha circondato le città di Peschici, di Vieste e che ha colpito il Gargano, nonché esprimere apprezzamento per lo sforzo della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, delle forze dell'ordine, della Guardia costiera, dei volontari, impegnati insieme alle autorità pugliesi e locali nello sforzo di vicinanza e di aiuto alle popolazioni colpite, molte delle quali sono delle popolazioni turistiche, che erano lì in vacanza.

Signor Presidente, cari colleghi, signor Ministro, desidero prima di tutto esprimere la solidarietà mia e del mio Partito al ministro D'Alema per l'inqualificabile attacco mediatico e giudiziario di cui è vittima in questi giorni. I suoi comportamenti possono essere oggetto di censura politica, ma è una pessima abitudine italiana sostituire alla censura politica l'azione giudiziaria. La censura politica si esercita nelle Aule del Parlamento e non nei tribunali. Questo appartiene all'abc della separazione dei poteri, teorizzata da Montesquieu alle origini dello Stato moderno e dello Stato di diritto.

magistratura e politica. Spiace dover rilevare che in altre, analoghe, circostanze, altri Capi dello Stato non hanno avuto uguale determinazione nel difendere le ragioni della Costituzione italiana. Spiace dover rilevare che, in occasioni analoghe, altre opposizioni non hanno avuto eguale senso dello Stato. Veniamo ora alla relazione. Signor Ministro, esistono cose che condividiamo e altre che non condividiamo. Le dirò subito che la cosa che ci ha più colpito è stata l'ultima, l'idea di una politica estera per la pace. Questa è un'idea che ha animato la politica estera italiana dopo la fine della Seconda guerra mondiale ed è l'eredità più alta che, da De Gasperi ad Andreotti, la fase democristiana della storia del Paese lascia a quelli che hanno successivamente esercitato responsabilità di Governo: una politica per la pace. Su questo non possiamo non sottolineare con forza il nostro accordo. Tuttavia, una politica per la pace richiede una visione ampia, di lungo respiro; una politica per la pace interviene prima che i conflitti siano così esacerbati da aver fatto scorrere il sangue. Su questo avremmo gradito sentire qualcosa in una visione di sviluppo dell'area mediterranea, dove molti conflitti stanno fermentando e che oggi, con una politica di pace, possono essere fermati; una politica di pace una politica preventiva della guerra, una politica che sa investire. Non è un uso di parole per sottrarsi a responsabilità, per non incorrere in spese e in rischi. È un modo di spendere e di rischiare prima, per prevenire la guerra. Penso all'Algeria, alla Tunisia, penso a tutto il Mediterraneo occidentale. Credo che su questo sarebbe necessario avviare una riflessione più approfondita. Francamente, non abbiamo trovato nella sua relazione respiro strategico: i soldati italiani sono sparsi per il mondo in missioni di pace, ma lei non ci ha spiegato perché. Avrei gradito ascoltare qualcosa sulla minaccia che il terrorismo oggi rappresenta per le società libere nel mondo; avrei gradito vedere inquadrati questi interventi all'interno di una lotta contro il terrorismo, che stiamo conducendo insieme con i nostri alleati e avrei gradito anche sentire richiamare quello che è sempre stato il punto fermo della politica estera italiana, l'amicizia con gli Stati Uniti, ulteriormente rafforzata dal quadro della Alleanza Atlantica. *(Applausi dei senatori non è giusto dire che nel passato l'Italia ha consumato sicurezza. No! L'Italia ha prodotto sicurezza; l'ha prodotta per sé, per i Paesi vicini, per il mondo intero, attraverso le scelte illuminate di De Gasperi, che ci ha fatto aderire all'Alleanza Atlantica e ci ha fatto creare la Comunità Economica Europea. Questi sono stati i due pilastri della politica di pace dell'Italia. Allora, la politica di pace aveva anche chiarezza nell'individuare gli avversari perché la pace è minacciata e bisogna chiamare per nome chi minaccia la pace: ieri l'impero sovietico; l'altro ieri il nazifascismo, oggi il terrorismo e, in modo particolare, il terrorismo islamico, che sta lanciando una grande offensiva in tutto il mondo contro i regimi liberi, non solo contro le società occidentali, ma anche contro i Paesi islamici moderati. Fuori da questo quadro è assai difficile vedere le linee della politica estera di un grande Paese. Come giudicare Hamas, fuori del quadro della politica generale, volta a difendere la libertà contro le minacce attuali, fuori della lotta contro il terrorismo? Questo, mi spiace dirlo, non l'ho sentito. Non so se altri, all'interno dell'Aula lo abbiano sentito. Avremmo, inoltre, gradito sentir ricordare che perno della politica estera dell'Italia, dal punto di vista dei contenuti l'alleanza con gli Stati Uniti è un mezzo di politica estera - sono la difesa della pace ma anche la difesa della libertà. La difesa della pace e la difesa della libertà non possono essere separate. E difesa della libertà oggi è anche, forse e soprattutto, difesa della libertà religiosa. Oggi, nel mondo, la persecuzione contro i cristiani è la minaccia più grande, più evidente, più sanguinosa contro la libertà. Abbiamo vissuto di recente il caso drammatico di Padre Bossi. Ma lei sa quali sono le condizioni nelle quali operano i missionari italiani in tutto il mondo? Lei sa quali sono le condizioni di persecuzione nelle quali vivono i cristiani in un gran numero di Paesi? Non è questa una priorità per la politica estera italiana? Accanto ai cristiani, voglio naturalmente ricordare tutti coloro che sono perseguitati per la loro religione e, più in generale, per le loro idee. Può un grande Paese come l'Italia avere una politica estera in cui questa non è riconosciuta come una priorità? Eppure, nel suo intervento, di questo non abbiamo trovato menzione. Signor Ministro, mi consenta un'altra osservazione. Noi siamo impegnati nel Libano: qual è il quadro all'interno del quale comprendiamo il nostro impegno il Libano e anche gli sforzi che lei meritoriamente sta compiendo per la pace in Palestina? Anche qui c'è una parola che avremmo desiderato sentire e non abbiamo sentito. Noi crediamo che l'Italia e l'Europa abbiano l'obbligo morale di garantire la vita dello Stato di Israele all'interno di confini sicuri, internazionalmente riconosciuti. Vogliamo uno Stato palestinese, ma riteniamo che vada garantita la sicurezza dello Stato di Israele. Lei ha accennato ad errori che gli israeliani hanno commesso. Concordo con lei: gli israeliani hanno fatto molti errori. Ma sa qual è la radice di questi errori?

del mondo arabo voglia portare a compimento l'Olocausto. La paura è cattiva consigliera e fa commettere degli errori, ma Israele non sbaglia ad avere paura, perché esistono nel mondo arabo forze potenti che vogliono completare l'Olocausto. Quelle forze vanno condannate, non sono oggetto di un dialogo possibile: su che cosa trattiamo con queste forze? Di non far fuori tutti gli israeliani, ma magari solo uno sì e uno no, o uno su dieci? Ci Ci sono questioni sulle quali bisogna avere il coraggio di prendere posizioni forti e decise, sulle quali bisogna avere anche il coraggio di accettare lo scontro. Il diritto di Israele alla vita non è oggetto alla vita non è oggetto di trattativa, nemmeno con partiti che avessero eventualmente forte radicamento democratico. Le ricorderò che molte rivoluzioni, nate con l'appoggio democratico, sono poi terminate nel sangue e nell'oppressione. Possiamo riconoscere come interlocutori Governi i quali ritengono di non avere un dovere di rispetto del diritto di Israele all'esistenza? Infine, vorrei rivolgere un appello ai senatori a vita. Molto si è discusso sul loro ruolo. Io vorrei dire loro: votate pure la mozione del Governo, ma se non voterete la nostra mozione, quella firmata dai Capigruppo dell'opposizione, dovrete spiegarcelo; questo gesto o avrà una ragione di contenuto forte o apparirà come l'obbedienza ad un ordine di scuderia, la rinuncia a quell'indipendenza di giudizio di cui voi dovete essere i primi rappresentanti all'interno di questo Senato. Io vi invito ad agire e a valutare secondo coscienza la la mozione del Governo, ma anche quella che noi abbiamo proposto; mi sembra difficile immaginare una sola ragione per la quale voi possiate non votarla. Se agirete così, così, darete prestigio a questo Senato e a voi stessi, e rivendicherete i migliori valori e la continuità di una politica estera che alcuni di voi hanno meritoriamente condiviso a costruire.

il signor Ministro per la vasta e stimolante relazione che ha dato un po' il quadro del pianeta e della nostra situazione all'interno di questo mondo complesso. Immersa in un'estenuante battaglia tutta concentrata sui fatti, grandi, piccoli e anche inesistenti della politica interna italiana, quest'Aula si è assai poco applicata ad analizzare un mondo sempre in costante trasformazione. Questo credo sia un segnale di conservatorismo e anche una manchevolezza. È ovvio che in questo mio intervento non è possibile trattare della complessità del globo; rimarrò quindi all'interno dei parametri tracciati, toccando alcuni punti focali. Con la costante crescita sia demografica che economica di un buon numero di Paesi in Asia e in America latina, è normale che l'Italia riduca il proprio peso relativo nello scacchiere internazionale e che debba, con audacia e intelligenza, ridisegnare il proprio profilo. È chiaro che gran parte del destino del nostro Paese è legato all'Unione Europea. Tuttavia, una politica di dogmatismo neoliberale della Banca centrale europea e un allargamento troppo rapido della frontiera nella ricerca di aree di nuova colonizzazione verso Est, che ci costringe ad ingoiare Governi come quello dei gemelli Kaczynski in Polonia, ci porta all'impossibilità di promuovere una politica estera e di difesa comune. Una parte considerevole di tale incapacità europea deriva dalla sottomissione militare agli Stati Uniti e dalla permanenza in una struttura superata come quella della NATO. Dal momento che l'Italia è una media potenza e inoltre sta perdendo forze in termini relativi, non possiamo accusarla dei mali del pianeta: ciò è ovvio. Ma, d'altra parte, essa non può neppure intromettersi in missioni militari, tentando di risolvere problemi al di là di quanto le sue forze permettano, e quelle alle quali partecipiamo già sono troppe. vi sono questioni che obbligano qualunque uomo o donna con responsabilità di Governo a tentare di dare il proprio contributo. Fra di essi, il più clamoroso è il dramma di quel minuto pezzo di terra che chiamiamo Israele e Palestina. È da sei decenni che si dichiara che due popoli devono coesistere in due Stati, e tutto tende a peggiorare. Signor Ministro, devo dire che apprezziamo molto la lettera, sebbene timida, dei dieci Ministri degli esteri europei, della quale lei è stato uno dei redattori, consegnata a Tony Blair, nuovo inviato del Quartetto per il Medioriente. Personalmente, considero la designazione di Tony Blair una bestemmia, ma questo è un problema diverso. Nella lettera i Ministri tendono a ristabilire il diritto internazionale, avendo come obiettivo una pace fra i Paesi dell'area, senza esclusioni, la garanzia della sicurezza per tutti, un cammino per la costruzione di uno Stato palestinese e la denuclearizzazione della Regione. Credo sia corretta, direi che è quasi ovvia, la posizione che si debba dialogare con tutte le parti rappresentative in causa, e questo include Hamas. Non riesco a capire come si possa raggiungere la pace fra avversari armati e contrapposti senza negoziare, ascoltare, tentare di capire la posizione di tutte le componenti. La guerra al terrorismo, intercalata dal bombardamento delle popolazioni civili in diverse zone del pianeta, portata avanti in primo luogo dall'amministrazione di George W. Bush *junior*, non ha solo causato dolori, distrutto corpi e anime, aperto le porte dell'inferno, ma è stata anche controproducente rispetto ai fini dei suoi autori. Meno di un mese fa, i servizi di sicurezza statunitensi divulgavano un rapporto dal titolo «Al Qaeda meglio organizzata per colpire l'Occidente». Bel risultato se dopo sei anni assassini come quelli di Al Qaeda si diffondono in decine di Paesi, sono stelle televisive e polo di attrazione per migliaia di islamici takfiristi! Al contrario, l'esempio di un'efficace politica di pace è quella della missione UNIFIL nel Sud del Libano, al momento sotto il comando del generale di divisione Claudio Graziano. Dobbiamo lamentare la morte di diversi caschi blu, spagnoli e colombiani: ad essi e alle loro famiglie va il nostro pensiero ed il ringraziamento per il compito che hanno svolto. Lì però la pace è stata mantenuta, i terreni sostanzialmente sono stati sminati e la popolazione apprezza l'intervento. Non credo che si possa dire lo stesso dei popoli che abitano lo spazio afgano. Centinaia di civili sono stati sterminati nelle ultime settimane dai bombardamenti della NATO e degli Stati Uniti. I diritti civili non si estendono, ma le coltivazioni del papavero da oppio sì. È necessario riconoscere che le missioni non funzionano e scavano vieppiù l'abisso già esistente tra l'Occidente e le altre culture. Ad ottobre l'Italia dovrà presentare all'ONU la relazione sulla missione militare in Afghanistan. È con la massima serietà che noi le chiediamo, signor Ministro, di proporre che la missione militare passi nelle mani dell'ONU, e solamente dell'ONU, con una forza di *peacekeeping*, con l'obiettivo di proteggere la popolazione civile. Insisto e sottolineo che per il nostro Gruppo tale questione è essenziale. essere che l'Italia non abbia la forza per modificare il carattere della missione, ma in tale caso non vediamo perché continuare con la nostra presenza militare. Infine, vi è un'altra situazione che guardiamo con molta preoccupazione. Il Governo degli Stati Uniti d'America ha già affermato di essere pronto a riconoscere una dichiarazione unilaterale di indipendenza della regione autonoma del Kosovo. Questa gravissima violazione della risoluzione 1244 dell'ONU calpesterebbe, una volta di più, il diritto internazionale e riaprirebbe le ferite ancora bagnate di sangue nei Balcani, mentre la probabilità di nuovi conflitti in Bosnia e, più al Sud, fra serbi e albanesi, sarebbe molto alta: tutte aree nelle quali si trovano dislocati distaccamenti consistenti di nostre truppe. Non dubito che il Governo italiano avrà una posizione di massima responsabilità e accortezza, ben sapendo che non esiste soluzione che non sia condivisa anche dalla Serbia. Per concludere, voglio ancora rendere esplicita la nostra ferma opposizione a qualsiasi partecipazione diretta o indiretta dell'Italia al cosiddetto progetto di «scudo stellare» che, per il momento, coinvolge la Repubblica Ceca e la Polonia. Questo potrebbe riaprire, nelle nuove condizioni, un capitolo che pensavamo chiuso per sempre, quello della guerra fredda, cosa che non possiamo permetterci per gli attuali popoli d'Europa e per le sue future generazioni. Una meravigliosa notizia sarebbe, invece, che il Governo italiano decidesse, una volta per tutte, di bloccare le minacce di concedere un ampliamento della base «Dal Molin» a Vicenza. Certamente, ciò rafforzerebbe la pace in Europa e la salute dell'attuale Governo. La ringrazio, signor Ministro, e le auguro

tant'è che il suo intervento si qualifica come relazione in materia di politica estera, con particolare riferimento alle operazioni di pace.

La legge dice: «Il Governo riferirà». Mi sarebbe piaciuto che il Ministro della difesa fosse al suo fianco oggi, e che entrambi riferiste in Aula.

sulla contrarietà da parte dell'estrema sinistra alle operazioni di pace e alla politica estera in generale, tanto è una litania che sto sentendo da un sacco di tempo. Alla fine, se costoro saranno effettivamente contrari alla politica estera

contrario, vuol dire che sono solo capaci di reiterare azioni criminose come quelle che stanotte sono state perpetrate nei confronti

durerà in eterno e quali sono le prospettive di soluzione politica. Venga il Governo a riferire quali sono le prospettive di soluzione politica, quali iniziative sul piano politico intende adottare.

forze, sul Kosovo, in termini di quadro di situazione e di prospettive, però, mi scusi, non ha detto una parola sulla Bosnia né, soprattutto, sull'Afghanistan. Perché? L'Afghanistan non è forse un discorso terribilmente impegnativo per le nostre operazioni?

Non ho sentito alcun riferimento sullo sforzo di partecipazione ad iniziative per la lotta al terrorismo in ambito europeo. Sarebbe opportuno che ci si rendesse conto che la principale minaccia nei confronti dell'Unione europea è rappresentata dal terrorismo. So di non scoprire niente di importante, lo ripetiamo, ma vorrei sapere cosa si fa, in termini unitari, comunitari, per preparare le forze, integrare, scambiare l'*intelligence* nei confronti di questa minaccia.

assai interessanti che lei ha detto, relative specificatamente alla politica estera, parlerà il collega Mantica in sede di dichiarazione di voto*.* Quello che ci attendiamo è che vi sia una partecipazione integrata del Governo, e non del Ministro degli affari esteri da una parte e del Ministro della difesa dall'altra; che siano indicate le prospettive politiche, e non soltanto la realtà riferita alla situazione che serve: bisogna dire quali sono le prospettive;

Poi che ci dica quali sono le iniziative di Governo nei confronti delle situazioni di crisi che riguardano la minaccia alla sicurezza mondiale, dove noi siamo...

puntualissimo. La conclusione è la seguente. Cerchiamo di realizzare una politica estera unitaria, cerchiamo di presentarci in Parlamento uniti e non divisi. Noi di Alleanza nazionale auspichiamo che anche nell'ambito della compagine governativa - che non ci è certamente molto simpatica - si trovi una unione, una integrazione perfetta,

e starei per dire quasi completa. Dico "quasi" perché mi sembra che ci siano della lacune, benché in molti settori, come quello, per esempio, dell'Europa, lei sia stato molto dettagliato. Nell'insieme, direi che la sua relazione mostra una grande volontà politica positiva, che trovo molto apprezzabile, che è di riuscire ad avere almeno la fede, la speranza di poter risolvere, avviare a soluzione o migliorare le condizioni di qualsiasi area di conflitto attraverso forme di dialogo. Purtroppo, però, sappiamo bene che il dialogo da solo non produce nulla, in mancanza di una strategia globale e, come già è stato detto da altri colleghi, con tutto il rispetto, devo dire, e l'ammirazione per la sua complessa relazione, non sono riuscito a scorgere una strategia globale di politica estera che non vada al di là di una enunciazione di atti dovuti e apprezzabili e di enunciazioni anch'esse apprezzabili, ma che non portano da sole da nessuna parte. Che cosa mi ha colpito di più? È stata, ad esempio, l'assoluta mancanza del tema dell'Iran. Lei ha parlato della moratoria della pena di morte, lodevole proposito, ma la moratoria della pena di morte ha dei soggetti. Ora io non so se anche il suo *computer*, onorevole Ministro degli affari esteri, ma certamente il mio e quello di molti altri ricevono ogni giorno filmati raccapriccianti su esecuzioni pubbliche che avvengono quotidianamente e più volte al giorno, nelle piazze e nelle strade dell'Iran: esecuzioni di minori; esecuzioni che avvengono per impiccagione attraverso delle gru mobili oppure attraverso la lapidazione che viene compiuta scavando la buca e mettendo il condannato dentro alla buca fino alla testa, con

della frattura palestinese. Non basta dire che bisogna auspicare una ripresa di rapporti fra Hamas e Al Fatah: questa ripresa di rapporti non ci sarà mai, non è possibile, perché Hamas ha come riferimento l'Iran; Hezbollah ha come riferimento l'Iran; la Siria, in cui succedono anche cose positive, per quella parte invece che resta legata al traffico delle armi e alla paralisi dello sviluppo del processo libanese dipende dell'Iran; l'Iran oggi governa di fatto una larga parte dell'Iraq

Allora, non possiamo omettere questi elementi dello scacchiere. Come pure, d'altra parte, non possiamo non ricordare che la situazione di Gaza non capita a caso;

una questione umanitaria gravissima. Gaza era una delle zone più fiorenti ed è stata data ai palestinesi

distrutta, polverizzata da quella parte del popolo palestinese che non vuole assolutamente alcuna pace, non vuole procedere in alcun modo ad alcun riconoscimento di Israele, né oggi né mai, e con la quale il presidente Abu Mazen ha detto che non ci sarà mai alcun dialogo (e non ci deve essere alcun dialogo). Allora mi chiedo: come queste lacune? C'è un'altra lacuna che trovo importante. Capisco che, se parlo del caso Litvinienko, molti potranno pensare che ne parlo anche per fatto personale: è vero, è un mio fatto personale, ma la guerra fredda che molti paventano ha purtroppo delle venature di attualità e c'è una crisi diplomatica profonda tra il Regno Unito e la Federazione russa, con l'espulsione di diplomatici. In questa situazione si è inserita anche l'Amministrazione americana, con una dichiarazione molto forte di Condoleezza Rice, e Sarkozy è l'unico presidente dell'Europa continentale che abbia saputo esprimere al nuovo Governo di Gordon Brown la propria solidarietà nel momento in cui il Regno Unito l'ha chiesta e nessuno altro Paese, tranne, appunto, la Francia di Sarkozy, l'ha concessa. Dove eravamo noi? Dove siamo noi? Da che parte siamo noi? Queste sono domande non provocatorie, ma che riguardano problemi attuali e reali, ai quali certamente va risposto non in maniera arrogante, non in maniera muscolare, anzi bisogna mostrare sempre l'intelligenza,

bisogna essere tutti buoni, bisogna che tutti dialoghino, bisogna creare delle agenzie internazionali e svilupparle affinché possa intercorrere questo dialogo, e così via; certamente,

eurasico sono gravi e importanti perché mostrano anche un problema strategico - che lei, signor Ministro, conosce bene - tra le due vocazioni dell'Europa: quella quella euro-asiatica, che coincide anche con il sogno gollista e con molti altri sogni, e quella di un'Europa *partner* atlantico. All'epoca del giovane Gorbaciov, quando assunse il potere, la sua posizione era abbracciare l'Europa, mettendo fuori gli Stati Uniti. Una parte dell'Europa oggi continua a perseguire lo stesso fine. Non c'è nulla di male, a parte che detesto questo fine; però, è un problema che va affrontato:

agli Urali e chiude a lucchetto sulla Manica e sull'Atlantico o è un'Europa anche ampia ad Est, ma che non chiude nulla ad Ovest e che, anzi, comprende al suo interno la fondamentale amicizia con la più la più grande democrazia del mondo, insieme alla madre di tutte le democrazie, che è appunto il Regno Unito? Non si può essere strabici o stare con un piede di qua e uno di là, mentre i due continenti si divaricano e si finisce per terra. Non basta dire che bisogna essere

ed anche apprezzabili; ma esse sono totalmente mancanti di una strategia e sembrano - mi perdoni l'espressione - un po' un minestrone, specie se diluite in un tempo piuttosto lungo. Guardavo poi la reazione che ha suscitato il suo discorso a sinistra; lei avrà notato che l'estrema sinistra dello schieramento politico che sostiene il suo Governo è rimasta gelida e impassibile e non l'ha applaudita, con poca generosità. Questo dimostra, a parere mio, che anche la sua relazione, signor Ministro degli affari esteri, risente delle gravissime spaccature e conflittuali divisioni che esistono all'interno della sua maggioranza, che la sua relazione purtroppo, malgrado i grandi e buoni elementi che contiene, non poteva non riflettere.

dalla costruzione europea ai recenti sviluppi nel Consiglio europeo, alla nostra iniziativa sulla moratoria della pena di morte alle Nazioni Unite, all'azione dell'Italia in ambito multilaterale del G8, alla posizione del nostro Paese sullo *status* finale del Kosovo. Considerazioni da noi pienamente condivise. Concentrerò la mia attenzione sulle missioni internazionali nelle quali il nostro Paese è impegnato in aree di vitale interesse strategico nazionale e anche in altre nelle quali il nostro Paese è chiamato a dare un suo proprio contributo nella lotta al terrorismo e in ragione del suo ruolo nella comunità internazionale. infatti, partecipa a numerose missioni internazionali, mantenendo fuori area quasi 10.000 dei nostri soldati, per il mantenimento e la promozione della pace, sotto l'egida delle Nazioni Unite, della NATO, dell'Unione Europea. Lo fa con coerenza, con capacità, con orgoglio, con onore. Oggi il nostro Paese è particolarmente impegnato con i suoi contingenti militari, oltre che nella ex Jugoslavia, in Afghanistan e nel Libano, dimostrando grande affidabilità e capacità professionali e operative che ne hanno accresciuto il riconoscimento e il prestigio nel mondo. A tutti i nostri soldati rivolgiamo il nostro saluto, il nostro apprezzamento, il nostro grazie per il loro impegno e il loro sacrificio nella difesa dell'interesse nazionale. Nei riguardi dello scacchiere mediorientale l'onorevole Ministro ha ricordato i risultati della recente conferenza di Roma sull'Afghanistan, sottolineando l'importanza di promuovere e sostenere la creazione in quel Paese di un vero Stato di diritto. Egli ha anche ribadito l'importanza del dispiegamento militare UNIFIL in Libano, che va considerato uno snodo fondamentale per la sicurezza di tutta la regione. Condividiamo questa valutazione dell'onorevole Ministro; non sottaciamo tuttavia - a differenza di come fa egli stesso - la difficile situazione in Afghanistan anche per i nostri soldati, che ha richiesto, tra l'altro, un rafforzamento delle attrezzature militari a loro disposizione, e dove i progressi per il controllo del territorio sono scarsi, nonostante le azioni militari NATO intraprese specie nel Sud-Est del Paese, che hanno purtroppo causato anche numerose vittime civili. È pur vero che l'opera di ricostruzione civile e di aiuto allo sviluppo, condotta dalla comunità internazionale e dall'Italia, continua senza sosta e comprende la riabilitazione di strade, la fornitura di acqua, la riapertura delle scuole, l'assistenza medica alla popolazione e l'economia dà segni di ripresa, anche se i problemi rimangono immensi. In Libano sono sorti nuovi rischi per la sicurezza del Paese dagli attacchi contro le forze militari libanesi di formazioni fondamentaliste, come Fatah al-Islam, che potrebbero coinvolgere anche il contingente UNIFIL, come è successo con l'uccisione dei sei soldati spagnoli e colombiani, a seguito dell'esplosione di mine piazzate su strade da essi pattugliate. L'onorevole Ministro ha anche sottolineato il massimo impegno del nostro Paese per il rafforzamento del Governo Siniora. Ma al riguardo sarebbe importante per il Libano che le varie forze politiche in campo trovassero un accordo presto sulla personalità cristiano-maronita da eleggere questo autunno come nuovo Presidente della Repubblica, e ricercassero ogni intesa necessaria per dare al Paese un Governo di unità nazionale. Su questi due fronti, Afghanistan e Libano, pertanto, nonostante i rischi, l'Italia deve rimanere impegnata con i propri contingenti militari, continuando al contempo a svolgere la più intensa azione diplomatica nella ricerca di soluzioni durature e pacifiche. Appare chiaro, però, che in questi teatri non bastano la presenza e l'azione militare; sono necessarie - lo ripeto - nuove iniziative politiche, senza le quali anche la tregua in Libano, alla quale hanno contribuito con successo UNIFIL e il nostro contingente, non potrà durare. Il ministro D'Alema ha ricordato il recente incontro sul Libano organizzato dalla Francia a La Celle Saint Cloud, al quale hanno partecipato anche rappresentanti di Hezbollah. Benché non sia stata raggiunta l'intesa su un documento politico conclusivo, credo che tale incontro, tale dialogo sia stato utile. L'Italia, dati i suoi buoni rapporti con tutti i Paesi dell'area mediorientale, è ben qualificata a portare avanti nuove iniziative diplomatiche per ricercare soluzioni condivise e risolvere le tensioni e i conflitti in atto. Sul fronte israelo-palestinese, l'aspro conflitto fra le due forze politiche palestinesi, conclusosi con la piena presa di controllo della striscia di Gaza da parte di Hamas e con la fine del Governo di unità nazionale con Al Fatah, ha prodotto un tale deterioramento del quadro politico in Palestina che oggi mancano i presupposti politici minimi per riavviare il dialogo fra le forze politiche; ma a questo non ci dobbiamo rassegnare. In queste circostanze, condividiamo la posizione del nostro Governo (come quella del Consiglio dei Ministri degli esteri dell'Unione Europea), di ferma condanna per il colpo militare di Hamas e di sostegno che dobbiamo dare al nuovo Governo di Al Fatah, guidato da Salam Fayad e dal presidente Abu Abbas. Governo italiano che ha incoraggiato il dialogo bilaterale con Israele e il rilascio di 250 prigionieri palestinesi detenuti in Israele stesso. Sono stati annunciati anche sostanziali aiuti economici al nuovo Governo palestinese da parte degli Stati Uniti, oltre all'annuncio, da parte del presidente Bush, di una conferenza internazionale nella prospettiva di creare uno Stato palestinese che abbia continuità territoriale. Ho notato con soddisfazione che il nostro Governo intende impegnarsi particolarmente per favorire la partecipazione a tale conferenza, prevista per il prossimo settembre, anche dei Paesi arabi, inclusi quelli che non hanno relazioni con Israele, come l'Arabia Saudita. Nel frattempo, è importante evitare una crisi umanitaria a Gaza, dove la situazione si sta avvicinando al collasso economico e ad una ulteriore radicalizzazione politica. È indispensabile che Al Fatah ricerchi appena possibile l'apertura di un dialogo con Hamas che auspicabilmente conduca a una riconciliazione, necessaria per condurre nel tempo alla creazione di uno Stato palestinese. È vero che Hamas è tuttora definita una formazione terroristica che non riconosce l'esistenza di Israele, ma è anche vero che Hamas ha vinto elezioni democratiche in Palestina, elezioni volute in particolare dagli Stati Uniti. La vittoria su Al Fatah è stata principalmente una reazione alla corruzione che è esistita nel Governo palestinese. Aprire un dialogo con Hamas non significa negoziare direttamente con Hamas, come ha detto l'onorevole Ministro. La partecipazione di Hamas a negoziati politici non è possibile fino a quando Hamas stessa non riconoscerà il diritto di Israele ad esistere come Stato indipendente entro confini sicuri e garantiti. Tuttavia, è utile rivolgere un incoraggiamento ad Abu Abbas con l'aiuto dei Paesi limitrofi a ricercare una riconciliazione fra i palestinesi. Onorevole ministro, le rivolgo, a nome del nostro Gruppo, tutto il nostro apprezzamento e i migliori auguri per la sua azione condotta nell'interesse del Paese.

vorrei fargli notare, con un po' di sorpresa e di tristezza, la freddezza e il distacco che ha mostrato nei confronti di Israele. Israele ha tre ostaggi di cui non abbiamo parlato mai: tre giovani soldati di cui non sappiamo nulla e sui quali non è mai stata fornita alcuna indicazione in alcun modo. Ancora ricordo i volti delle madri, dei padri e dei fratelli che si sono presentati alla nostra Commissione affari esteri per chiedere che facessimo qualcosa per loro. Israele ha due nemici: Hezbollah e Hamas, a Nord e a Sud, due tra le organizzazioni più

un impegno di guerra. Lei, signor Ministro, ha parlato di errori riferendosi unicamente ad Israele: mi pare che l'area sia molto più drammatica e che forse l'occasione di oggi ci avrebbe consentito di ricordare che quel Paese ha appena eletto Presidente della Repubblica un Premio Nobel per la pace e una grande personalità del socialismo internazionale: Shimon Peres. Mi permetta, a nome di quest'Aula,

sarò molto breve perché ho illustrato ciò che dovevo in una relazione molto lunga e d'altro canto credo che, innanzi tutto, il Governo debba registrare i suggerimenti e le osservazioni del Parlamento e tenerne conto nello sviluppo del nostro lavoro. Io vorrei chiarire, dato che diversi colleghi hanno obiettato l'assenza di un disegno strategico, che naturalmente il Governo ha presentato le dichiarazioni programmatiche. In occasione della nascita del Governo, io ho presentato alle Commissioni di Camera e Senato un'ampia relazione sulle strategie della politica estera, dove venivano richiamati i princìpi e i cardini della politica estera italiana. Ora, sinceramente, non credo che sarebbe ragionevole che ogni sei mesi, quando la legge ci chiede di fare il punto sulle missioni internazionali, io venga qui a riesporre la strategia della politica estera italiana. mi sono limitato a fare il punto sulle principali questioni di politica estera che sono nell'agenda internazionale, riferendomi in modo puntuale a ciò di cui si è discusso a giugno e a luglio e a ciò che è in agenda tra settembre e dicembre. Naturalmente, è del tutto evidente che questo approccio è parziale, non comprende un esame di tantissime questioni, ma è esattamente il punto sulla politica estera italiana, non l'illustrazione di una strategia che certamente avrebbe richiesto di discutere delle relazioni transatlantiche, della nostra visione dell'Asia e di tantissimi altri problemi di cui non ho parlato. ho parlato. L'orientamento del Governo, però, è noto, fa parte delle dichiarazioni programmatiche e ad esse rinvio chi abbia dei dubbi circa il fatto che abbiamo deciso di abbandonare le tradizionali alleanze del nostro Paese, Paese, dubbi, naturalmente, infondati. Vorrei dire al senatore Buttiglione, che ringrazio, innanzi tutto, per le espressioni di solidarietà che ha voluto esprimere verso di me, da autentico garantista qual è, è, che ha sollevato un tema effettivamente cruciale, e cioè la lotta contro il terrorismo. In effetti, se non del tutto, tuttavia in una parte notevole, l'impegno internazionale del nostro Paese in missione di pace è collegato al grande tema della lotta al terrorismo, ma è esattamente intorno a questo tema che si è sviluppato e si sviluppa una parte importante del dibattito internazionale a cui noi ci riferiamo. cioè, non è se lottare o meno contro il terrorismo; il problema che si è posto a noi, all'intera comunità internazionale e, in primo luogo, al sistema politico e all'opinione pubblica degli Stati Uniti è se la strategia della guerra al terrore, che si è manifestata in modo particolare nella decisione di una guerra preventiva e unilaterale nei confronti dell'Iraq, si sia rivelata una strategia efficace. Ed è proprio qui, mi permetto di dire, che noi abbiamo cercato di avviare un corso di politica estera volto a contribuire - perché naturalmente l'Italia da sola non lo potrebbe fare - a voltare pagina rispetto ad una stagione nella quale l'idea di fermare il terrorismo con la guerra si è rivelata controproducente sotto il profilo del terrorismo che, semmai, come dicono oggi gli stessi servizi americani, ha accresciuto la sua pericolosità e ha portato ad una grave divisione del mondo occidentale, innanzi tutto tra una parte consistente dell'Europa e gli Stati Uniti d'America. ha reso drammatico il confronto tra mondo occidentale e gran parte del mondo islamico, quando invece è chiaro che la condizione fondamentale per sconfiggere il terrorismo è costruire una coalizione in grado di coinvolgere tanta parte del mondo islamico, perché il terrorismo non è nemico dell'Occidente, è nemico dell'umanità ed è innanzitutto nemico di ogni aspirazione di progresso e di modernità all'interno del mondo musulmano ed arabo. Ed è esattamente a questo mutamento di orizzonte che il Governo italiano ha cercato di contribuire, con una politica che ha messo l'accento sul multilateralismo e sulla costruzione di una vasta coalizione internazionale, anziché sulla logica di tipo unilaterale. Si può essere d'accordo oppure no con questo sforzo, ma esso è esattamente un'ispirazione politica e non semplicemente una dichiarazione di buona volontà. Ripeto, è un'ispirazione politica che ha cercato nel corso di questi mesi di rimettere in campo l'azione delle Nazioni Unite, come è avvenuto nel Libano, di rilanciare l'idea di un'azione comune dell'Europa e non di una *coalition of the willings*, e che ha cercato ovviamente di rilanciare il dialogo con gli Stati Uniti in questa prospettiva. Siamo, infatti, ben consapevoli che l'unica possibilità perché questa politica abbia successo è che ad essa partecipino gli Stati Uniti, anche sotto l'impulso di un'opinione pubblica americana che largamente chiede un mutamento di politica estera. Questo è il contesto: lo si può non condividere, ma non mi sembra giusto dire che il Governo non abbia una sua ispirazione strategica. Poi, Poi, naturalmente, dentro questo contesto: si collocano le singole questioni che affrontiamo e il modo come cerchiamo di portare avanti le risposte.

B: abbiamo voluto oggi fare una discussione di politica estera perché questo era il desiderio espresso dal Parlamento. La legge non impone al Governo di venire in Aula e di votare ogni sei mesi sulle missioni, impone di informare il Parlamento, il che lo si può fare anche informando le Commissioni e non necessariamente l'Aula. Se siamo venuti in Aula è perché si è chiesto di avere un dibattito sulla politica estera e, se il Governo ha scelto che poi ci sia anche in Commissione - che non è una serie B del Parlamento, ma un suo organo un'informazione specifica sugli aspetti militari, è per offrire al Parlamento una maggiore ricchezza di informazioni e non certamente perché consideriamo la politica della difesa un aspetto secondario. un aspetto secondario. Non riprendo ciò che ho detto sull'Afghanistan, perché ne ho parlato, innanzitutto illustrando le conclusioni della conferenza che si è tenuta a Roma sulla giustizia, sulla *rule of law*, ma anche in relazione al difficile passaggio nel quale certamente è essenziale l'opera di sostegno alla formazione di istituzioni democratiche, di Forze armate e di una Polizia funzionante, perché lo scopo che abbiamo, in definitiva, non è quello di permanere in Afghanistan per un tempo indefinito, ma di aiutare quel Paese a camminare sulle sue gambe nel tempo più rapido possibile, anche se certamente non sarà un tempo breve. Vorrei dire una parola su un tema che evidentemente tocca sensibilità: questione israelo-palestinese. Non so se o come si possa misurare il calore delle parole; in generale, nell'analisi della politica estera cerco di essere freddo. Non credo che l'analisi che si fa in Aula della politica estera debba accompagnarsi ad espressioni di calore. Non c'è alcun dubbio che l'Italia concorra alla difesa della sicurezza di Israele e del diritto alla sua esistenza *(Applausi dal Gruppo Ulivo)* e che lo faccia non con le parole, ma con la forza degli atti e delle scelte politiche. Non a caso, il Governo israeliano ci ha espresso una grande gratitudine per avere dispiegato le nostre forze armate a protezione della sicurezza di Israele. E non vi è il minimo dubbio che, se nel momento attuale di drammatica tensione sul fronte palestinese, palestinese, invece di esserci l'UNIFIL ed i soldati italiani ci fosse Hezbollah al di là della linea di confine, oggi Israele sarebbe infinitamente meno sicuro.

E penso che si è amici di Israele, se lo si incoraggia e lo si aiuta a perseguire la via della pace, con i palestinesi e con l'insieme del mondo arabo. Il che richiede una azione politica

Non voglio entrare ora in una analisi (che, tuttavia, forma oggetto di un vasto dibattito internazionale) sulla natura di Hamas e sulle possibili prospettive di evoluzione di questo movimento e sulla natura di Hezbollah**,** che è altra cosa, in quanto non è presente in nessuna lista di movimenti terroristici. Fa parte del Parlamento libanese ed ha fatto parte del Governo fino a qualche mese fa, ma questo dibattito è aperto, innanzitutto, in Israele.

senza le prevenzioni ideologiche che imprigionano il nostro dibattito, credo che potremmo, con molta serenità, cercare di vedere qual è la via più conveniente per arrivare alla pace. Torno a dire che sono colpito

di quel Governo Sarkozy che in altre sedi è indicato come un modello della destra europea e che, se prende una iniziativa per il Medio Oriente, invece, diventa paraterrorista, salvo arrivare un po' grottescamente a rappresentare, come qualcuno ha fatto su qualche organo di informazione, la lettera del Ministro degli esteri dell'Europa mediterranea come un'iniziativa di D'Alema, il quale non era neppure presente alla riunione in cui è stata concordata, anche se la condivide. Pertanto, abbiamo una sorta di destra europea *à la carte* che quando serve diventa un modello, ma quando prende iniziative che non sono utili alla polemica di politica interna viene messa al bando. Trovo singolare che questa iniziativa, che ha trovato nel Parlamento europeo un così largo sostegno, con una mozione che ha tra i firmatari l'onorevole Moscardini, Alleanza Alleanza Nazionale, i capi del Partito popolare europeo e che è stata approvata all'unanimità, debba diventare qui - permettetemi di dirlo - per ragioni di politica interna, un discrimine tra maggioranza e opposizione. Trovo che è proprio così che si finisce per trasformare anche la politica estera, anziché in una sede di confronto, in una palestra di polemiche esclusivamente legate al quadro politico nazionale. Secondo me è un errore e mi permetto di dirlo con grande serenità a persone che rispetto - alcune delle quali sono state anche protagoniste della politica estera italiana e che sanno benissimo che ciò che dico è tutt'altro che privo di fondamento. Detto questo, il Governo ringrazia il Senato: è stata una discussione utile e certamente terremo conto del contributo del Parlamento nello sviluppo dell'azione politica impegnativa che ci attende. apre una nuova finestra"). Prima di dare di nuovo la parola al Ministro per il parere sulle risoluzioni presentate, che sono tredici,

la Presidenza ricorda che il dibattito odierno si collega alla richiesta formulata dal senatore Calderoli e dai Capigruppo dell'opposizione il 9 luglio scorso, in relazione allo stato delle missioni internazionali,

nelle successive riunioni della Conferenza dei Capigruppo, la portata del dibattito è stata estesa alla politica estera, con particolare riguardo alle missioni internazionali. In questi termini ha disposto il calendario dei lavori dell'Assemblea approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, e conseguentemente è stato formulato l'ordine del giorno della seduta odierna. I contenuti delle proposte di risoluzione debbono quindi muoversi in tale ambito. Le questioni relative all'ampliamento della base di Vicenza sono state oggetto di mozioni discusse in Assemblea il 1° febbraio scorso, alla presenza del ministro Parisi. Successivamente, con dichiarazioni rese alla Camera dei deputati il 20 giugno, il Presidente del Consiglio ha dichiarato che le decisioni sulla base di Vicenza sono state già assunte ed ha confermato l'impegno del Governo. Per utilità, vi leggo le affermazioni del Presidente del Consiglio

ha infatti deciso di confermare una decisione già assunta dal nostro Paese con atti politici e amministrativi adottati dal Governo precedente e ratificati dalle autorità le stesse che - lo ricordo - sono state confermate alla guida del territorio vicentino in occasione delle recenti consultazioni amministrative. Il rispetto degli impegni presi è alla base del diritto internazionale e dei rapporti di pacifica convivenza tra i Paesi,

Come di consueto, le rimanenti proposte di risoluzione saranno messe ai voti secondo l'ordine di presentazione, una dopo l'altra. L'approvazione o la reiezione di ciascuna di esse non produrrà effetti di assorbimento né di preclusione.

che essa di per sé non reca un indirizzo di politica estera, ma riguarda le conseguenze, sul piano della continuità del Governo, di un eventuale voto del Senato nel quale fosse determinante il voto dei senatori a vita; sotto questo aspetto la proposta sarebbe estranea all'argomento all'ordine del giorno. In secondo luogo, la proposta riguarda un eventuale carattere determinante del voto dei senatori a vita. In questo modo essa pone una questione squisitamente istituzionale: pretende cioè di distinguere il significato e l'efficacia del voto dei senatori a vita da quello dei senatori eletti, ed introduce così una differenziazione nel corpo omogeneo del Senato che - come la Presidenza ha più volte avuto l'occasione di affermare e come ribadisce con fermezza anche nel caso presente - non ha alcun fondamento né nella Costituzione, né nel Regolamento della nostra Assemblea. Per tali ragioni, la proposta di risoluzione n. 9 è inammissibile.

argomenti che dovrebbero essere rispettati, fra cui anche la vicenda relativa alla caserma di Vicenza. Tengo a ricordarle ciò proprio perché è stato aggiunto, nella riformulazione, che a Vicenza è di stanza la 173ª Brigata,

Lei giustamente ricorda che il Parlamento si è già espresso in diverse sedute su tale argomento, ma non è colpa dell'opposizione, che ha presentato di risoluzione, se vi è una sottoscrizione di 170 parlamentari della maggioranza in cui invece si chiede una moratoria dello stesso. A fronte di numeri così consistenti della maggioranza, credo che il Parlamento debba decidere se questa moratoria debba esserci o meno. Sicuramente non avremmo ribadito l'impegno se qualcuno non avesse sottoscritto tale richiesta di moratoria, fra cui numerosi senatori.

sulla base di Vicenza. In occasione della Conferenza dei Capigruppo, avevo manifestato la mia estrema contrarietà alla sua prossima decisione. Lei si avvale del Regolamento e dei suoi poteri. Noi li rispettiamo, ma le segnaliamo che non condividiamo, perché riteniamo che lei stia consumando una strappo delle regole.

alla luce di questi fatti, abbiamo chiesto un dibattito sul contenuto dell'incontro avvenuto tra il Presidente del Consiglio e il Presidente degli Stati Uniti, contenuto che disconosciamo per il semplice motivo che il Ministro degli esteri non ce ne ha parlato. nasceva la nostra richiesta, che si è poi congiunta con quella del collega Calderoli, che chiedeva che il Governo riferisse in Parlamento

ed ecco che noi riteniamo e continuiamo a ritenere che si stia facendo uno strappo, perché questo tema attiene ad un dibattito di politica estera e perché così è calendarizzato e così risulta dall'espressione utilizzata per indicare l'oggetto dell'ordine del giorno.

ha dovuto subire, purtroppo per lui, la caduta del Governo; un'Aula che fa paura, tra l'altro, al nuovo emergente *leader* del Partito Democratico che, mezz'ora fa, ha dichiarato

prendiamo atto del fatto che la maggioranza non è in grado di discutere di Vicenza, perché discutendo di Vicenza si divide. Oggi ha deciso di non dividersi, vuole andare in vacanza senza mostrare divisioni: siamo rammaricati che il Presidente del Senato offra alla maggioranza, per così dire, lo strumento tecnico per non dividersi. Non si illudano, però: il problema rimane! Capiamo che il regolamento di conti verrà in autunno su un insieme di temi, tra cui le pensioni e l'Afghanistan (ho letto il documento sull'Afghanistan ed è incredibile quanto propongono 41 colleghi). Prendiamo atto che questa maggioranza non può reggere su nessuno degli argomenti fondamentali sui quali deve essere unita. Vuole andare in vacanza come Governo balneare? Vada pure! È un Governo balneare che va in vacanza. Pertanto, Presidente, consideriamo la sua decisione un aiuto alla maggioranza in un momento di difficoltà.

che siano state ritenute inammissibili le proposte di risoluzione aventi ad oggetto la vicenda relativa alla base di Vicenza, trova un principio di contraddizione nella stessa organizzazione complessiva dei lavori del Senato. I colleghi ricordano benissimo che quando si è discusso della base di Vicenza era presente

con la presenza del ministro Parisi per ragionare, appunto, delle comunicazioni del Governo sulla base di Vicenza. Ciò dimostra, ancora una volta, che questo argomento è estraneo a questo Consesso. Lo dico per capirci. Che poi la maggioranza non sia in nessun modo, come dire, disponibile a discutere dei temi di politica estera che possono essere considerati, e talvolta lo sono stati, elementi che hanno introdotto - com'è assolutamente normale nelle grandi coalizioni, in tutti Paesi del mondo - delle divisioni è dato dal fatto che oggi discutiamo di politica estera in quest'Aula e votiamo delle proposte di risoluzione credo per la settima volta.

ma sono totalmente in dissenso con la sua decisione e con la volontà dei Capigruppo che l'ha ispirata. La ritengo un errore,

da Vicenza sono partite le operazioni dei paracadutisti e delle forze aerotrasportate americane, sia per l'Iraq che per l'Afghanistan. Mi sembra quindi che si abbia paura di qualcosa di cui né il Governo, né, tanto

Se non voto contro la mozione della maggioranza, è proprio perché cerco di restare freddo e, forse, perché so che altri, non il sottoscritto, lavorano per indebolire questo Governo. Se mi astengo dalla votazione, sarà per fare dispetto a questi

Signor Presidente, capisco che sia un momento particolarmente difficile, ma vorrei riprendere una frase del ministro D'Alema e fare una battuta: capisco che la politica estera italiana ha un difetto, che difficilmente è estera, nel senso che molto spesso guarda a casa nostra. La decisione apparentemente regolamentare che lei ci ha comunicato è un classico atto di politica interna. Qui non si tratta di discutere sulla base di Vicenza, che è assolutamente congruente con il dibattito che stiamo facendo. C'è una posizione e mi spiace che la Presidenza del Senato si faccia carico di un problema della maggioranza, che forse riguarda più l'Afghanistan che la base di Vicenza e che attraverso un fatto regolamentare si impedisca a quest'Assemblea di esprimere liberamente un'opinione. un'opinione. Quando riceviamo lezioni dal Ministro su alcune posizioni che assume l'opposizione in quest'Aula, vorrei ricordare che la Presidenza del Senato, in questo caso,

Non è così. La gestione diretta della questione se l'è formalmente assunta il Presidente del Consiglio che, un mese fa, ha ribadito chiaramente la posizione del Governo. Non ne dobbiamo riparlare oggi.

Calderoli, siamo in una democrazia parlamentare, nella quale, se lei vuole interrogare il Governo sulla base di Vicenza può presentare un'interrogazione o un'interpellanza. Così funzionano le

Grazie, non l'avevo sentito.

perché esprime un giudizio pesantemente negativo rispetto all'iniziativa intrapresa dai Paesi europei dell'Europa mediterranea, sottoscritta anche dal nostro Governo e quindi è in palese contrasto con le comunicazioni che ho fornito qui, che hanno invece ribadito i valori di questa iniziativa e hanno ricordato come essa sia stata apprezzata dal Parlamento europeo.

Per quanto attiene alla seconda affermazione, che appare leggermente contorta, tuttavia mi sembra evidente che riferendosi agli impegni assunti dall'Italia nelle missioni internazionali i supporti logistici sono quelli delle Forze armate italiane e noi siamo a favore della logistica delle Forze armate italiane.

si profila complesso e lungo ed è volto a costruire la pace e la stabilità, sulla base di quanto ho illustrato al Parlamento. Questo

il Governo esprime un parere favorevole: al di là di formulazioni che appaiono discutibili, ma la sostanza del dispositivo è che si impegna il Governo ad un ruolo propulsivo per la pace, per il disarmo nucleare (che è esattamente uno tema sul quale ci stiamo impegnando); l'abbandono delle guerre preventive è un appello superfluo perché noi siamo contrari, l'abbiamo dimostrato ritirando le nostre Forze armate dall'Iraq, tuttavia *ad abundantiam*;

Tra l'altro, introduce la percezione che la NATO sia impegnata sul territorio iracheno, il che non è vero, perché la NATO è presente soltanto con una missione di *training* che si svolge a Baghdad e non su tutto il territorio iracheno. iracheno. Sinceramente rischia di determinare confusione, non mi sembra accoglibile per il modo in cui è formulata. dal senatore Calderoli, contiene considerazioni polemiche verso singole personalità della maggioranza, eccetera, che a mia giudizio hanno poco a che fare con con il dibattito di politica estera e il Governo esprime un parere contrario; tanto più che la parte positiva di questa proposta di ribadire il valore del rapporto con gli Stati Uniti mi pare assorbito dal parere favorevole sulla precedente proposta di risoluzione che va in questo senso. La proposta

La premessa mi sembra inutilmente polemica verso colleghi che sono qui e con i quali si può discutere senza questi *escamotage*. Il parere favorevole, quindi, è limitato al dispositivo. il parere è negativo perché conferma tutte le missioni internazionali avviate nella scorsa legislatura e non potremmo votare a favore avendo ritirato le Forze armate dall'Iraq quindi, avendo agito in un senso diverso rispetto a quello auspicato dalla proposta di risoluzione. Per quanto riguarda la proposta di questa non è accoglibile perché il Governo intende partecipare alla Conferenza intergovernativa sulla base del mandato approvato dal Consiglio europeo, del mandato approvato dal Consiglio europeo, che non prevede una correzione del Preambolo. Quindi, noi saremmo incoerenti con la volontà di partecipare alla conferenza allo scopo di realizzare il mandato deciso dal Consiglio europeo. Siccome ci sono altri Governi, come quello della Polonia, che vogliono riaprire la discussione, se anche noi ci mettessimo su questo piano, creeremmo - credo - un grave danno alla prospettiva di quell'accordo faticoso che è stato raggiunto e che ora bisogna semplicemente tradurre in un nuovo trattato.

Mi è rimasta la facoltà di ritirare

È chiaro che ogni documento contiene tanti apprezzamenti e tante frasi condivisibili, ma sinceramente questo esercizio di spezzettare i concetti non mi sembra che alla fine produca una sintesi perspicua, nel senso che quello che decide il Senato deve essere comprensibile all'opinione pubblica. Quindi, do atto a tutte le proposte di risoluzione di contenere tanti riferimenti positivi; però, il giudizio si volge complessivamente ad accogliere quelle che sono accoglibili e non a spezzettare tutte le altre per togliere i riferimenti che non convincono, altrimenti qui saremmo impegnati in un lavoro di macelleria delle proposte di risoluzione che durerebbe giorni e giorni

cancellando questi due righi, visto che tutto il resto è esattamente la questione sulla quale chiediamo al Governo un'opinione. D'ALEMA,

senatore Castelli,

e consideri seriamente le frasi, gli incisi, i punti, le virgole ed i punti e virgola: infatti, sa benissimo - al par di me e di tutti coloro che sono qui - che in queste proposte

«ad operare in stretta cooperazione con tutte le Forze NATO impegnate in altre aree del territorio iracheno nello sforzo di costruzione della sicurezza interna irachena, premessa indispensabile di stabilità di governo».

è accaduto che, a commento della sua decisione, il collega Calderoli citasse esplicitamente il Capo dello Stato

È chiaro che se l'opposizione intende espungere dalle risoluzioni tutti i riferimenti critici al Governo, questo le approverà e ringrazierà l'opposizione. Potrei fornire una lista completa, per

Signor Presidente, signor Ministro, mi occorre pochissimo tempo per dire che i senatori e le senatrici dell'Italia dei Valori sosterranno la proposta di risoluzione di maggioranza. Da un po' di tempo in quest'Aula dibattiamo di politica estera forse in modo più frequente rispetto a quanto sia giusto fare, però, da un anno a questa parte, noi ritroviamo una continuità nella politica estera della nostra Nazione - mi spiego - rispetto a quella che è stata la politica estera dell'Italia dal dopoguerra in poi. Una continuità che si ritrova sui valori dell'atlantismo, sui valori fondanti delle Nazioni Unite, una continuità che ci consente di poter dire che oggi noi pratichiamo, così come per il passato, una politica filo‑occidentale attenta ed autonoma. Questo è quello che ci piace segnalare rispetto a ciò che era avvenuto in precedenza. La nostra politica filo-occidentale attenta ed automa si contrappone invece ad una politica filo-occidentale non attenta e non autonoma che aveva caratterizzato la legislatura precedente. precedente. Se il nostro Ministro degli affari esteri oggi può dire, così come ha detto, che fermare il terrorismo con la guerra è stato controproducente, io penso che possa farlo perché noi siamo autonomi e attenti a quel che avviene complessivamente nell'ambito delle alleanze che nel Patto atlantico e sulle Nazioni Unite fondano la loro solidarietà. Concludo quindi confermando il voto a sostegno della proposta di risoluzione di maggioranza dei senatori e delle senatrici dell'Italia dei Valori.

a nome dei senatori del Gruppo della Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia la solidarietà al ministro D'Alema, come agli altri colleghi che ne sono stati oggetto, per l'attacco mediatico - giudiziario attacco che ripropone il delicato problema di un corretto rapporto tra organi giudiziari e rappresentanze istituzionali e che ogni giorno di più è evidente nel nostro Paese. Detto questo, i senatori del nostro Gruppo non voteranno per la proposta di risoluzione di maggioranza e voteranno invece a favore delle diverse risoluzioni presentate dai senatori Schifani, Pianetta, Mantica, Marini Marini e Calderoli. Non possiamo votare la proposta di risoluzione che approva le comunicazioni del Governo non per un preconcetto di opposizione ma perché le dichiarazioni del Ministro degli esteri, pur contenendo considerazioni sulla politica europea e sull'impegno italiano per l'abolizione della pena di morte su cui conveniamo e su cui vasto è il consenso di tutte le forze politiche, appaiono, per altri versi, assai contraddittorie. In particolare pur riconoscendo, a proposito della missione UNIFIL, il permanere di infiltrazioni di armi dalla Siria al Libano e il fatto che il controllo dei confini libanesi è oggi insufficiente, ci è apparso che, sul punto, egli sottovaluti i pericoli e la gravità della situazione. Basta ricordare le dichiarazioni al quotidiano in lingua araba «Hayat» dello sceicco Mohammed Yazbek, membro dell'ufficio politico di Hezbollah, che ha affermato: «Rispetto alla guerra dello scorso anno le nostre capacità sono quasi raddoppiate, siamo pronti ad ogni eventualità. Se il nemico si è preparato ed è pronto, noi pure siamo pronti a impartirgli una lezione che non dimenticherà». La dichiarazione, arrivata dopo l'incontro a Damasco tra il segretario generale degli Hezbollah, Nasrallah, con il presidente Ahmadinejad e con quello siriano Bashar al‑Assad, è resa più significativa dal ruolo che lo sceicco Yazbek ricopre, cioè quello di rappresentante ufficiale in Libano della guida suprema iraniana, l'ayatollah Khamenei. Ci saremmo quindi aspettati dal Ministro alcune precise proposte da avanzare in sede di Nazioni Unite sul come rendere più incisiva la missione UNIFIL e non solo l'affermazione che, secondo il capo del Governo libanese, è necessario estenderla sino al 2008. Del pari, pur ribadendo l'importanza della Conferenza tenuta a Roma sull'Afghanistan, ella, onorevole Ministro, ha piuttosto posto l'enfasi sulla necessità di un confronto internazionale, promosso dall'Italia sul valore della missione afgana. Forse perché era condizionato dall'appello firmato da 41 senatori della sua maggioranza proprio questa mattina, che hanno affermato: "attendiamo ancora la svolta in Afghanistan. La coalizione internazionale sembrerebbe aver rinunciato a praticare una netta discontinuità rispetto al passato. Per queste ragioni torniamo oggi a chiedere al Governo italiano di impegnarsi per un'effettiva inversione di rotta". Proseguivano poi in questo appello, dichiarando che "la soluzione diplomatica dovrà essere perseguita con massima determinazione attraverso una conferenza internazionale, coinvolgendo l'Europa, i Paesi presenti con propri contingenti militari e i Paesi confinanti, nonché tutte le componenti del popolo afgano, chi accetta la presenza delle truppe internazionali e chi la osteggia". Quindi, secondo questi colleghi, anche i talebani. su questo punto delicato, se il Ministro avesse voluto precisare una posizione chiara, evidentemente avrebbe determinato non pochi contrasti Per quanto riguarda il problema dei rapporti israeliano‑palestinesi, ci è sembrato che ella abbia voluto oggi correggere le sue precedenti dichiarazioni di San Miniato, ribadendo il ruolo di Abu Mazen e la sua personale amicizia con lui. Tuttavia, francamente, questo non ci appare ancora sufficiente. Hamas è un'organizzazione che ha un programma di guerra, di terrorismo e di distruzione di Israele. Non riteniamo possa mai essere coinvolta in un processo di pace, di costruzione dello Stato palestinese, se non ripudia il terrorismo come strumento di lotta e non accetta di riconoscere il diritto all'esistenza di Israele. Ogni pur cauta apertura, di credito, verso questa organizzazione, il permetterle di ritenere che vi possa essere nei suoi confronti un ammorbidimento della comunità internazionale, senza che essa modifichi le sue posizioni, è qualcosa che non rafforza Abu Mazen e non avvicina il processo di pace in quella martoriata area. Negli scorsi giorni - credo l'abbia ribadito anche poc'anzi in Aula - un autorevole collega della sua parte politica, il senatore Furio Colombo, ha scritto su «l'Unità» "è chiaro a tutti ormai che senza Israele non ci sarebbe mai stata neppure la rivendicazione di uno Stato palestinese, dal momento che Giordania ed Egitto si erano già attribuite parte del territorio che avrebbe dovuto diventare Palestina". E proseguiva, affermando che "senza la permanenza stabile e sicura di Israele e del suo diritto alla pace non ci sarà mai alcuna patria dei palestinesi, ma soltanto guerriglia senza fine". Sono affermazioni che condividiamo totalmente. La difesa del diritto di Israele ad uno Stato sicuro, secondo il Gruppo dei senatori della Democrazia cristiana, del Partito repubblicano, del Movimento per le autonomie, deve rimanere il punto centrale di ogni politica italiana nel Medioriente. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, credo che l'occasione per dibattere sulla politica estera sia sempre un momento di grande rilievo per il Parlamento italiano, per le nostre istituzioni, ma, soprattutto, per la nostra politica. Credo che nella relazione del Ministro degli esteri ci siano stati sicuramente - come ricordava il collega Buttiglione

alla sicurezza e tanti riferimenti anche del Governo, sull'azione della Farnesina, sulla politica estera nel nostro Paese, ma, soprattutto, anche il riferimento alla coerenza di una politica estera che intende essere sottolineata anche in quest'Aula.

di valutare argomenti importanti come il tema del Mediterraneo e le priorità italiane che da sempre sono la vocazione naturale della nostra politica estera e che segnano il passo io credo in questi ultimi anni: le politiche del Mediterraneo, la politica dei Balcani, dell'America latina, tutti argomenti che ritengo sostanzialmente importanti, come quello della cooperazione culturale, che troppe volte è rimasto assente. Abbiamo ricordato, noi per primi, dell'UDC, che la cooperazione culturale deve servire a far capire nel mondo che l'Italia è una superpotenza non militare, ma culturale e la diplomazia preventiva, alla quale il collega Rocco Buttiglione ha fatto riferimento, la grande rete politica, culturale, di solidarietà nella quale deve rimanere impigliata la pace è la politica che noi di ispirazione cristiana, che usiamo lo stesso linguaggio dei cittadini, non solo italiani, europei e del mondo, vogliamo rappresentare anche in questo contesto. E proprio per questo anche io vorrei ripetere l'appello

se lei rappresenta, con la sua politica, una autorevole posizione personale o se la sua politica la rappresenta anche il suo Governo, la sua maggioranza. Noi abbiamo una visione romantica della politica estera. Pensiamo che la politica estera di un Paese rappresenti il luogo naturale, dove si saldano i valori condivisi della comunità nazionale, si fissano le priorità. E qui non ho ascoltato priorità, ho ascoltato un elenco di problemi importanti. Su queste priorità, con le quali ci si apre al confronto con le altre realtà nazionali e sovranazionali, ci si sente accomunati da un comune destino e sorretti da un'unica conoscenza ed identità. Questa è la politica estera che noi immaginiamo, che tra l'altro lei ha accennato, la politica estera dell'Italia, se davvero vuole essere condivisione di valori, come molti colleghi hanno accennato in Aula, e coscienza matura dell'intera nazione non può prescindere da alcuni princìpi indefettibili:

signor Ministro degli esteri. Ma la credibilità non può derivare da un esercizio acrobatico, come ho visto fare anche nell'Aula, nell'espressione dei pareri; un esercizio acrobatico che non sta nella qualità di eccellenza anche della sua figura, signor Ministro, che noi rispettiamo. E non pensiamo assolutamente che le sue dichiarazioni siano in libertà

la ricomposizione delle lacerazioni, delle divisioni, delle contraddizioni che alcuni colleghi della maggioranza hanno evidenziato in modo coraggioso, di una maggioranza politica, quale essa sia, perché la credibilità di una politica estera non può prescindere, a mio parere, da una ricerca costante di una condivisione allargata a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, nella consapevolezza che il destino di una maggioranza non possa rappresentare il destino del Paese. Proprio per parlare del tema principale, quello che ci ha portato a discutere, voglio ritornare sulla questione di Hamas, tramite il suo *leader*, che ha ringraziato il ministro D'Alema per le sue parole. Lo ha fatto in maniera convinta e noi vogliamo sottolineare senza acredine questa posizione politica.

con Abu Mazen, ha parlato di amicizia con il *Premier*; è uno strano modo di essere amici quello di affermare che Hamas è una forza reale di rappresentanza e che rappresenta gran parte del popolo palestinese. Signor Ministro, pensiamo che lei noi sia uno sprovveduto, ma una persona da stimare, perché nella diversità delle impostazioni ha il coraggio di fare delle dichiarazioni, ma è nostro dovere sottolineare le differenze, le differenze, anche con quella che noi pensiamo dovrebbe essere l'iniziativa dell'Italia. L'iniziativa di D'Alema tende, a nostro parere, a legittimare con queste parole Hamas di fronte alla comunità internazionale. Con questa iniziativa del Ministro degli esteri italiano appare evidente che Hamas ha così segnato un punto nel braccio di ferro con il presidente Abu Mazen, la cui posta in gioco è il diritto di rappresentanza dei palestinesi. Appare evidente che il Ministro degli esteri voglia accettare come interlocutore gli integralisti di Hamas al posto del moderato Abu Mazen. Non ci convince nemmeno la teoria delle democratiche elezioni, che hanno legittimato Hamas. In quelle dichiarazioni noi non ci ritroviamo, ma siamo però d'accordo con l'ambasciatore israeliano Meir, il quale ha ragione quando ricorda al ministro D'Alema che anche Hitler vinse, come Hamas, democratiche elezioni e che quello non può essere un argomento buono per legittimare dei fanatici estremisti. Non è possibile. Lei ha fatto molti riferimenti a sintonie europee, o meglio, alla moderazione europea,

con le proprie illusioni, pensa di poter trattare con chiunque, anche con il diavolo, trovandosi comunque il tornaconto. È pura illusione a nostro parere pensare di negoziare con il fanatismo religioso nell'utopia di una reciproca soddisfazione. E allora, signor Presidente, noi registriamo che gli stessi francesi hanno preso le distanze dalle sue parole, da questa politica. Il ministro D'Alema è certamente coerente e questa coerenza vogliamo portare all'attenzione del nostro Parlamento. Su questa coerenza c'è continuità tra le diverse iniziative del Governo Prodi nello scenario del Medioriente. Infatti, ai tempi della guerra in Libano (luglio 2006) lo stesso ministro D'Alema legittimò gli Hezbollah con parole simili a quelle usate

degli Hezbollah e di Hamas, sono certamente coerenti e il senatore Guzzanti su questo tema ha detto delle cose che noi condividiamo. Consentitemi di dubitare che l'arrendevolezza nei confronti degli estremisti e dei loro *sponsor* serva alla stabilità del Medioriente e quindi agli interessi dell'Italia e dell'Europa. Credo che il Parlamento italiano il Senato della Repubblica possa trovare lo spazio per riconoscere che buttare a mare i moderati, come oggi Abu Mazen, e legittimare gli estremisti è sempre stata, tra tutte le politiche, la peggiore.

la relazione del ministro D'Alema, per la chiarezza di princìpi che l'ha ispirata, per la trasparenza degli obiettivi politici indicati ed anche per il realismo dell'analisi dei fatti. che proprio questo mi pare il punto fondamentale da recuperare insieme, in questa fase così difficile della politica internazionale, ossia il senso del limite della nostra politica estera come il senso della complessità del quadro dello scenario internazionale che stiamo vivendo e rispetto al quale non mi pare abbondino a livello internazionale ricette semplici.

sottolineando le presunte ambiguità della politica estera del Governo. Vedete, colleghi, noi viviamo una fase nella quale grandi e molteplici sono gli elementi di incertezza del quadro internazionale. Ciò non impedisce al nostro Governo e alla maggioranza che lo esprime di avere una chiarezza forte su quali siano gli obiettivi di fondo della nostra politica politica estera, che hanno fatto la storia della politica estera italiana dal dopoguerra ad oggi, potremmo dire da De Gasperi a Prodi. Innanzitutto, vi è la centralità della costruzione di un'Europa politica insieme e inscindibilmente con l'amicizia transatlantica con gli Stati Uniti e una forte politica mediterranea per la pace, politica mediterranea per la pace, resa ancora più interessante dal fatto che questo mare, che un tempo si chiamò "nostro", ai tempi dell'antica Roma, è tornato ad essere centrale nello scacchiere internazionale. Dopo essere stato marginalizzato, paradossalmente, dalla scoperta dell'America ad opera di un italiano, il Mediterraneo oggi è tornato ad essere un elemento centrale nei traffici mondiali ed è strategico per il nostro Paese lavorare per la pace nel Mediterraneo. Credo che il Parlamento sia unito su questi tre punti. Vorrei dire ai colleghi dell'opposizione che non è una grande politica presentare il Paese diviso, quando esso nella sua stragrande maggioranza - e questo Parlamento ne è perfettamente espressione

Su questi tre punti la politica estera italiana è unitaria e può vedere l'unità del Parlamento, delle forze politiche e del Paese. Dopodiché, ci sono i problemi di fronte ai quali ci troviamo e, in particolare, le tre aree nelle quali, tra l'altro, sono presenti le nostre truppe. Il ministro D'Alema, con grande onestà intellettuale e politica, le ha indicate come situazioni problematiche, che tali sono e tali restano.

da rendere difficile quella conquista delle menti e dei cuori che è l'elemento strategico per il successo del Governo Karzai. Ricordare questi fatti non è pusillanimità di fronte alla guerra al terrorismo, ma un elemento di realismo senza il quale la guerra al terrorismo diventa retorica che costruisce da sola la sua sconfitta. Dobbiamo invece lavorare affinché l'intervento in Afghanistan

sullo Stato di diritto, pur presentando elementi, se vogliamo, di forte volontarismo, certamente va in quella direzione, nella direzione giusta. Il secondo *dossier*

Chi può dire di avere la chiave per la soluzione di quel problema? Ci troviamo davvero di fronte ad un contesto nel quale facciamo i conti (pensiamo, ad esempio, alla vicenda che ha lacerato la comunità palestinese) con il grande dilemma del mondo arabo nel nostro tempo,

con tratti anche sanguinari in molti casi (pensiamo a cosa è stato il regime di Saddam Hussein in Iraq), che tuttavia garantivano una pace interna, naturalmente relativa e macchiata da crimini orrendi, dall'altra parte

l'alternativa al regime corrotto di Al Fatah, che ha provocato una giusta reazione da parte di tanti palestinesi, per finire naturalmente nel rischio di un Hamas che può essere lo strumento di una rivoluzione di totalitarismo fondamentalista? Questa è la tragedia nella quale vive il mondo arabo. Com'è possibile pensare ad una politica estera del nostro Paese che insista in quell'area senza fare i conti con questa tragedia? Allora, è evidente che il filo per noi non può che essere quello

E se c'è stata una gigantesca esibizione muscolare, è stata la guerra in Iraq, con quello che è costata in termini di risorse e di vittime, da una parte e dall'altra: abbiamo ereditato

Dico questo non per contrapporre argomento ad argomento, ma per dire che siamo davvero in un contesto di grande difficoltà e delicatezza. Credo allora che una politica condivisa, da parte nostra, sia una politica che faccia i conti con realismo con tale situazione, tenendo aperto quell'unico filo che ci può portare da qualche parte, tentando cioè di moltiplicare le occasioni di confronto e di dialogo per arrivare a quella soluzione di pace che tutti riteniamo l'unica giusta e quindi possibile nell'area, vale a dire il pieno riconoscimento dei diritti dello Stato di Israele, il diritto all'esistenza e a vivere in pace e in sicurezza e, dall'altra parte, il diritto del popolo palestinese ad avere un suo Stato e un suo Governo.

per mascherare quella che invece sarebbe una solidarietà interna del nostro Paese nella sua proiezione internazionale. Infine, il terzo *dossier*, non meno complesso e delicato, è relativo al Kosovo, Kosovo, poco evocato nel dibattito di oggi. Si tratta di un tema assolutamente delicato e difficile. Ho colto nelle parole del ministro D'Alema una realistica considerazione della debolezza della proposta europea avanzata dal mediatore Ahtisaari. Ne abbiamo parlato ampiamente anche in Commissione affari esteri del Senato. Certamente anche in quel caso ci troviamo di fronte ad una contraddizione tra la spinta forte, che viene in particolare dall'Amministrazione americana,

Non mi riferisco soltanto alle zone dove sono presenti contingenti militari italiani, ma anche alle condizioni conflittuali caratterizzanti buona parte dello scacchiere mondiale. In Europa siamo, di fatto, spettatori pressoché inerti di un processo di grave arretramento. Questo per quanto riguarda le ormai lontane ambizioni di riuscire a costruire una comunità, l'Unione Europea, in grado di pesare non esclusivamente sul piano economico e finanziario, ma su quello diplomatico e della sicurezza. L'euro è, da tempo, la moneta più forte del mondo, ma i suoi possessori, i popoli europei, pesano assai poco nella soluzione dei problemi mondiali e su quelli stessi del vecchio Continente. La preclusione britannica, fortificata dalla surreale opposizione polacca, ha avuto la meglio quanto alle prospettive di innovazione. Marchiamo il passo. L'Europa tarda ad essere quell'entità politica obiettivo minimo dei fondatori dell'Unione. dell'Unione. Al di là delle dispute sul ruolo della Commissione e del Consiglio, e sul loro funzionamento, si addensano nubi oscure che minacciano la sicurezza e la pace medesima in primo luogo qui, ai nostri confini. Per quanto gli albanesi non accettano un'autonomia che non sia anche totale indipendenza per quella terra solcata da secolari contrasti e da guerre feroci.

L'Italia, che con America, Russia e Francia fa parte del gruppo di contatto chiamato a trovare la difficilissima soluzione, deve impegnarsi a non accettare né avallare alcuna decisione unilaterale. deve impegnarsi a fondo, anche più degli altri, perché noi più di altri siamo coinvolti, non solo per la vicinanza territoriale e per la presenza di nostri militari nella zona, ma perché duramente provati nella nostra stessa coscienza nazionale dalla tragica guerra della NATO contro la Jugoslavia alla fine degli anni Novanta. Guardando all'Est del Continente, si scorgono pericoli non meno gravi, i missili russi puntati sulle capitali d'Europa in risposta all'installazione di armi ultrapotenti da parte degli americani ai confini della Russia: proprio lì, cioè obiettivamente contro la Russia e non contro gli improbabili missili iraniani. Dunque, sono armi puntate sull'Europa

L'Italia e l'Europa non possono stare a guardare. Certo, sono preoccupate ed allarmate ma, sostanzialmente, ignave. Le minacce di una politica aggressiva dell'Iran vanno fronteggiate con fermezza politica e mezzi diplomatici, coinvolgendo in una comune responsabilità Europa e Stati Uniti con i Paesi arabi. In questo si esprime il nocciolo della linea del Governo italiano per il Medio Oriente. Io condivido questa linea, condivido l'analisi e le indicazioni del ministro D'Alema, ben sapendo che, come egli ha ripetutamente sostenuto, l'origine degli incendi che hanno infuocato quelle regioni e quelle popolazioni sta nel non risolto problema palestinese, non risolto dopo mezzo secolo: cinquanta terribili anni. E senza la creazione dello Stato di Palestina, che è diritto inalienabile del popolo palestinese, lì non vi potrà essere sicurezza per nessuno. La sicurezza stessa d'Israele, che è diritto inalienabile di quel popolo, non potrà fondarsi all'infinito sulla forza dei suoi armamenti. La pace in tutta l'area nasce e sparisce a fasi alterne, perché è solo tregua. Pace si avrà soltanto nel riconoscimento e nella esistenza di due Stati per due popoli: la terra dei palestinesi deve tornare ai palestinesi tutta intera, determinando con questo che la sicurezza di Israele potrà essere sicuramente riconosciuta, sicuramente garantita. E dopo la drammatica scissione tra i palestinesi, vanno sostenuti gli sforzi per accelerare, non per allontanare il processo di pace. Questo sta facendo il Governo italiano, intervenendo politicamente verso il Governo d'Israele, verso il Governo di Abu Mazen, verso Siria e verso Iran, verso Libano, verso Egitto, verso i Paesi arabi e verso gli attuali governanti della Striscia di Gaza. La pace si costruisce con atti di pace. I pericoli sono gravi, ma più gravi sono i pericoli e più grandi devono essere gli sforzi di pace per coinvolgere tutti, per non isolare nessuno e quanti dal proprio isolamento possono trarre soltanto conclusioni e atteggiamenti di esasperazione certo gravi e da contrastare, ma pur sempre pericolosi e insidiosi. Con la guerra non si risolve nulla: non si risolve in Iraq, dove l'ostinazione aggressiva del Governo americano va incontro ad una inevitabile disfatta, mentre l'Europa, l'Unione Europea, come ha dimostrato proprio ieri Sergio Romano sul «Corriere della Sera», in Iraq è stata già sconfitta, e non si risolve in Afghanistan, dove l'occupazione militare non ha fatto progredire né la sicurezza, né lo sviluppo di quel popolo. Da quel territorio, signor Ministro, cari colleghi, è ormai giunto il momento di programmare seriamente il rientro dei nostri militari. Il voto del Gruppo Insieme con l'Unione, a favore della politica estera qui esposta dal ministro D'Alema, si accompagna al nostro impegno per tale obiettivo. il nostro Gruppo voterà a favore delle comunicazioni del Ministro degli affari esteri, di cui condivide molte affermazioni. Prima di tutto, il forte richiamo al ruolo dell'Europa nella politica estera, come fattore di stabilizzazione e di pace. Ed è proprio per questo che siamo preoccupati per l'abbandono progressivo della strategia del disarmo nel nostro Continente. Ne ha parlato anche Benedetto XVI, domenica Abbandono della strategia del disarmo che si sta realizzando attraverso gli Accordi bilaterali tra Stati Uniti, Polonia e Repubblica Ceca per impiantare in quei Paesi il sistema dello scudo spaziale, teoricamente in funzione anti-iraniana. Questo ha determinato reazioni molto aspre da parte della Russia, che lo ha giudicato una minaccia agli equilibri preesistenti, aumentando a sua volta una ripresa dell'*escalation* negli armamenti. Questo alimenta un clima di vera e propria guerra fredda. Non solo. La Russia, dopo aver offerto agli Stati Uniti, senza esito, l'alternativa di trasferire in Azerbaigian il sistema di difesa missilistica, ha deciso la moratoria dell'accordo CFE per il controllo delle armi convenzionali e ha dichiarato che se il dispiegamento del sistema antimissile in Polonia e nella Repubblica Ceca proseguirà, sarà costretta a sopprimere le minacce potenziali che vengono da questi dispiegamenti. Insomma, è un orizzonte minaccioso. È evidente che si è così determinata una tensione che due potenze extraeuropee - Stati Uniti e Russia - agitano sulla testa di un'Europa ancora debole politicamente e militarmente non autonoma, obiettivo ideale per un'azione destabilizzante della sua strategia. Giustamente lei, Ministro, ha giudicato inopportuno dal punto di vista del metodo questo accordo bilaterale su una materia che avrebbe dovuto essere trattata in sede multilaterale, per esempio in sede Nato. Il punto è che, parallelamente a questa Dichiarazione, l'Italia il 17 febbraio aveva già firmato un Accordo quadro bilaterale con gli Stati Uniti per la condivisione di tecnologia di difesa missilistica riguardante il sistema MBDS, appunto lo scudo antimissile. L'Accordo, che si è tentato di spacciare per mero scambio di informazioni o pura cooperazione tecnologica, anche se fosse autorizzato in ambito NATO, rappresenterebbe per il nostro Paese una scelta sciagurata, minacciosa e strategicamente destabilizzante. Abbiamo apprezzato, invece, le valutazioni espresse sulla necessità di impegnarsi

perché bonificare i bacini d'odio e consentire una vita più dignitosa per tutti, oltre che importante, è uno dei modi per prevenire l'attecchire di ideologie integraliste. Abbiamo anche condiviso le valutazioni sulla missione UNIFIL in Libano, di cui abbiamo apprezzato il fatto di essere avvenuta per impulso dell'Europa, decisa dall'ONU con il consenso dei belligeranti e che ha prodotto la sospensione delle ostilità. Si è creata la condizione per un processo di stabilizzazione che, anche se tarda ad arrivare (lei ne ha parlato tanto), va comunque perseguito con il coinvolgimento di tutti gli attori in campo, diretti ed indiretti dalla Giordania ai Paesi arabi). Siamo consapevoli che è una missione molto pericolosa e per questo credo che tutti in quest'Aula siamo molto vicini ai nostri soldati. Abbiamo anche apprezzato le sue posizioni equilibrate ed appassionate insieme nei confronti della difficile situazione in Palestina ed Israele e condividiamo il metodo della trattativa sempre, comunque e con chiunque. Anzi, il disastro politico e la mattanza umana del grande Medio Oriente (parlo di Afghanistan ed Iraq) è dovuto al fatto di avere trascurato la via della trattativa e di aver scelto la strada della forza e delle armi. Oggi anche negli Stati Uniti c'è un ripensamento rispetto al senso di queste guerre, non solo negli ambienti democratici e negli editoriali progressisti. Il politologo repubblicano Edward Luttwak ha scritto che per superare il senso di umiliazione e di sconfitta delle antiche nazioni del Medio Oriente - cito testualmente - occorre «evitare invasioni militari e lasciare che i popoli del Medio Oriente vivano la propria storia». Tradotto, significa che la strategia adottata fino adesso non ha pagato. Questo viene detto nello stesso momento in cui in Afghanistan la Nato giustifica le stragi "dal cielo" di civili affermando che questo succede perché le truppe di terra sono troppo scarse. In Afghanistan la Nato ha adottato comandi e metodi di «*Enduring freedom*»*,* confondendosi con essa, e questo rende il quadro sempre più drammatico. Che le truppe d'occupazione restino non e la soluzione del problema della sicurezza dell'Afghanistan, ma costituisce una parte del problema. Gli eserciti d'occupazione non hanno reso l'Afghanistan più sicuro e vivibile: c'è la corruzione che è aumentata, il narcotraffico, il dominio dei signori della guerra, l'insorgenza talebana. È una guerra di occupazione che ha peggiorato la situazione. Il nostro Paese resta in Afghanistan con i suoi militari, coinvolto in una guerra d'occupazione, non per migliorare le condizioni di vita degli afgani, che sono nonostante tutti i nostri sforzi peggiorate, come risulta dai tanti civili inermi ammazzati nei bombardamenti anche della Nato, ma in virtù anche della Nato, ma in virtù di una coalizione internazionale dominata dagli interessi geopolitici degli Stati Uniti. In questo modo il mezzo, la coalizione, diventa il fine. Il voto parlamentare sulla missione afgana lo scorso marzo fu dato - e anche per molti di noi della sinistra con una grande sofferenza - nella prospettiva di una svolta positiva che non si è ancora realizzata. Lei oggi ha parlato della Conferenza internazionale di pace; rimane un obiettivo condiviso, ma è importante riuscire a coinvolgere tutta l'Europa e tutte le organizzazioni internazionali e gli Stati Uniti al più presto. Questo non dipende solo da un fatto volontaristico. È importante farlo al più presto perché la pace in Afghanistan non è un problema anche della sinistra italiana o di tutta la maggioranza o di tutto il Parlamento, ma è un bisogno vitale per la popolazione afgana. Per questo occorre farlo in fretta.

Signor Presidente, una cosa di cui tutti siamo estremamente convinti è che il terrorismo oggi sia una minaccia e forse la prima minaccia mondiale cui noi dobbiamo prestare attenzione. I Paesi che hanno più mezzi, più disponibilità e che hanno conosciuto democrazie più solide hanno anche il dovere di farsi carico di neutralizzare i tentativi di destabilizzazione mondiale. Ministro, a noi poco importa come si chiamino i destabilizzatori. Siano Siano jihadisti, siano talebani, si chiamino Hamas piuttosto che Al Qaeda o Hezbollah, per noi sono una minaccia per l'umanità. Noi conosciamo un gravissimo reato: il crimine contro l'umanità; ebbene, questo si dovrebbe estendere dovrebbe estendere ad ogni atto di terrorismo, in quanto il terrorista o l'organizzazione terroristica non si pone il problema degli effetti che produrrà il proprio atto. il proprio atto. Il loro obiettivo può essere militare o può essere quello che può essere, ma se sulla loro strada si presentano uno, due, cento o civili inermi i terroristi non si fermano dal perseguire il proprio obiettivo; pertanto, va classificato come crimine contro l'umanità. Presidente, proprio perché questa è una lotta senza frontiere, noi come Paese civile, europeo ed occidentale non possiamo chiamarci fuori. Presidente, noi non possiamo nemmeno permettere che i nostri governanti, governanti, i nostri amministratori e i nostri referenti possano permettersi di andare in giro per il mondo a braccetto con chi appartiene ad organizzazioni terroristiche. Non possiamo nemmeno accontentarci e riconoscere queste organizzazioni dicendo che tutto sommato questi sono stati eletti democraticamente. Presidente, Hamas ha espulso tutti i rivali politici che aveva in Palestina, se non li ha arrotati o messi al muro, ma la giustificazione che voi date per poter mantenere contatti e rapporti è l'elezione democratica. mi spieghi una cosa allora: se Hamas si può riconoscere perché ha avuto un'investitura democratica, perché nei confronti della Lega il vostro partito non ha mai voluto dare dare la legittimazione? La Lega è sempre stato un partito non violento. Siamo sempre stati eletti democraticamente; l'unico errore che abbiamo fatto, secondo voi, è stato quello di voler non riconoscere uno Stato incapace di dare le risposte nel momento in cui vanno date, uno Stato che costa troppo, che è arcaico, che è inefficace e volerlo semplicemente sostituire con un Stato più moderno ad autonomie diffusissime, apprezzando il lavoro dei territori. In poche parole: non avete voluto accettare la Lega perché proponeva una cura semplicissima per il Paese che si chiama federalismo.

delle vostre caratteristiche, che sono più dettate o da opportunismo o da convenienza. Consentitemi di dire che il *leitmotiv* della sinistra, ancor prima che arrivasse l'illustre magistrato Di Pietro, era costituito dall'insindacabilità dei giudizi della magistratura, dall'indipendenza e dall'autonomia totale dei magistrati. Questo è valso fintanto che qualche magistrato non è venuto a scavare troppo vicino alle vostre proprietà e ai vostri orti; a quel punto, vi siete addirittura scagliati contro di preoccuparvi dell'importanza o della gravità costituzionale dello scatenare anche il Capo dello Stato contro alcuni magistrati non graditi per come operano nel frangente contingente.

politica estera e nei propri rapporti internazionali: parlare di discontinuità rappresenta un pericolo enorme per la credibilità del Paese che si sta rappresentando. Abbiamo capito di essere governati da un Governo sindacato-dipendente: come sapete, c'è chi è dipendente da tante sostanze; il nostro Governo, invece, è sindacato‑dipendente. Non si sarebbe mai potuta giustificare la riforma di un sistema che già non è sufficientemente garantista per le nuove e le future generazioni, soltanto perché non si sa contrapporre ai sindacati su richieste inconcepibili e anacronistiche per il momento e per la

lapidino le donne, concedano perfino la pena di morte ai minorenni, piuttosto che intervenire a fianco degli americani. Insomma, questo la dice lunga

Siamo a favore della pace, finalizzata però ad un contesto di pace fra Paesi, organizzazioni o Stati che si riconoscano reciprocamente. Non siamo disposti, invece, a trattare con chi apertamente dichiara di non voler rinunciare all'azione terroristica come strumento di lotta e che, del resto, non si riconosce reciprocamente, pur confinando sulle stesse terre.

esplosivi e via dicendo. A noi, signor ministro D'Alema, non basta che vengano assicurati alla giustizia i pochi responsabili o i docenti di questo tipo di scuola. Chiediamo che, anche per gli allievi, sia la giusta corresponsabilità. Con quale spirito queste persone, al momento non assolutamente toccate, possono permanere e collaborare con noi italiani? Li avevano addestrati

Signor Ministro, dice un proverbio Zen: «quando sei in cima alla montagna non smettere di scalarla». Nel nostro caso, che si tratti di seguire un cammino già tracciato, di esplorarne di nuovi o di mirare ad altre vette, la scelta non è tecnica ma politica. A volte si scelgono scorciatoie: è il caso del minitrattato europeo, per noi una sconfitta, giacché siamo convinti della necessità di una Costituzione europea democratica, frutto di un processo costituente dal basso, da affidare anzitutto a un'Assemblea costituente e ad un *referendum*. Continueremo pertanto a perseguire questo obiettivo, praticando la nostra scelta politica attorno ai grandi temi di pace, giustizia sociale, economica e ambientale, diritto al lavoro stabile e contrattualizzato e beni comuni. A volte si scelgono strade sbagliate, come la concessione della base «Dal Molin» agli Stati Uniti, una decisione che continueremo a contrastare con forte determinazione; altre volte si decide per la strada maestra - come lei ha fatto oggi - giustamente legando il tema dei mutamenti climatici, della povertà e dell'esclusione sociale ad un nuovo paradigma «civile» della sicurezza. Aggiungiamo che gli esiti del G8 di Heiligendamm dimostrano l'ipocrisia di quei governi il cui modello di sviluppo «energivoro» ed il sostegno a politiche liberiste continuano a produrre le cause prime dell'insicurezza. Pertanto, chiediamo a lei e al Governo italiano che sosteniamo, che il nostro Paese pratichi un nuovo approccio basato sull'equità globale, nel dopo Kyoto, per l'Africa e sulla questione cruciale che sarà oggetto della discussione del vertice euroafricano, degli accordi di partenariato economico che permetterebbero l'allargamento dei mercati per la UE a discapito delle prospettive di sviluppo sano per i Paesi *partner*. Le chiediamo fin d'ora di ripensare radicalmente la decisione di ospitare il G8 alla Maddalena nel 2009. Basta con i G8; pensiamo ad una formula che sia allargata, democratica e partecipata dai Governi e dai rappresentanti della società civile transnazionale. Anche questa è una scelta politica che riteniamo essenziale per costruire un Governo globale autenticamente multipolare e democratico. È una scelta condivisibile quella che lei oggi ha portato in quest'Aula, cioè di mettere al centro un approccio basato sui diritti umani, che oggi trova maggior espressione nella campagna per l'abolizione della pena di morte e nell'entrata del nostro Paese nel Consiglio ONU sui diritti umani. Orbene, ci sembra che questo Governo stia pazientemente costruendo la trama di un strategia a tutto campo per un nuovo concetto di sicurezza umana e di prevenzione civile e diplomatica dei conflitti e di contrasto al terrorismo internazionale. Lo fa attraverso il rilancio di strumenti di lotta alla povertà e cooperazione internazionale che, lungi dall'essere considerati ancillari rispetto allo strumento militare (noi ci batteremo affinché questo non contribuiranno a rafforzare le politiche di prevenzione dei conflitti e di costruzione delle condizioni sociali e culturali per la loro gestione e «metabolizzazione» nel tempo. Una cosa però è dire, l'altra il fare. Lei ci ha parlato di Afghanistan e vogliamo essere chiari: riteniamo che sia urgente una netta inversione di rotta. L'inasprirsi della situazione sul campo sembra indicare che non solo le modalità seguite per la ricostruzione e il *peacekeeping*, ma anche l'istituzione che si è incaricata di farlo (la NATO) stanno contribuendo a far precipitare il Paese nella guerra totale. Anche gli interventi negli altri settori previsti dall'*Afghanistan Compact*, incluso il programma giustizia, sembrano essere destinati a scarsi risultati. Per questo chiediamo maggior impegno per costruire le premesse per una soluzione negoziale che veda coinvolti e i Paesi confinanti. *(Brusìo).* PRESIDENTE. Scusi, senatore Martone, pregherei i colleghi di portare un po' di attenzione. È un dibattito importante

i Governi presenti in Afghanistan e il popolo afgano, chi sostiene e chi osteggia la presenza straniera. E pensiamo che il tempo a disposizione stia terminando. Ad ottobre lei andrà a riferire al Consiglio di Sicurezza ONU sulla missione ISAF e vorremmo che in quell'occasione si giochi la carta della Conferenza internazionale, e si debba chiedere la sostituzione del contingente ISAF con un contingente di polizia internazionale con mandato ONU. Ci ha poi parlato del Libano, Paese ora scosso dal nuovo conflitto aperto da Fatah al-Islam nei campi profughi palestinesi, brodo di coltura della disperazione di un popolo e dagli incerti esiti della questione relativa al tribunale per il caso Hariri. Quando si decise di inviare le truppe nella missione UNIFIL 2, si stabilì anche che tale fase sarebbe stata seguita da una fase negoziale e diplomatica di cui si è persa però traccia. Invece riemergono appelli una revisione del mandato UNIFIL 2, per renderlo più «aggressivo» e permettere il disarmo di Hezbollah. Una tale eventualità rischia, a nostro parere, di pregiudicare il processo di trasformazione di Hezbollah in forza politica, interlocutore per il processo di pace, certamente in una cornice di sicurezza garantita da UNIFIL e dal Governo Siniora. Dobbiamo evitare il ripetersi di quanto è successo con Hamas. Basta leggere le pagine del rapporto di fine missione dell'inviato speciale dell'ONU per il Quartetto, De Soto, per capire come il Quartetto, sotto pressione americana, non avesse alcuna intenzione di assicurare le condizioni per un'evoluzione politica di Hamas. Per questo condividiamo la sua preoccupazione circa la possibile marginalizzazione di Hamas e quella relativa al rischio di una intollerabile frammentazione della Palestina in due entità, con Gaza ridotta ad un *bantustan* sotto tutela armata. Crediamo che sia importante sostenere una Conferenza internazionale sul Medio Oriente, con un forte ruolo dell'Europa, dei Paesi dell'area e dell'Arabia Saudita *in primis*, che possa anche affrontare la questione dal punto di vista macroregionale. Per quanto riguarda il Kosovo, riteniamo che il rischio di una dichiarazione unilaterale di indipendenza, insieme allo stallo nella discussione dei Consigli di sicurezza, possano innescare una spirale incontrollabile di tensioni etniche e di violazione dei diritti delle comunità serbe. Pensiamo si debba insistere sul rafforzamento delle misure di costruzione del tessuto sociale interetnico, tutela delle minoranze e interventi nelle infrastrutture, nella scuola e nella sanità siano essenziali prima di pensare a qualsiasi ipotesi di assetto istituzionale. ha accennato al Darfur, seppur brevemente. Di recente l'UNDP ha parlato del Darfur come il primo conflitto scatenato dalla competizione su risorse naturali scarse, come l'acqua, conseguenza dei mutamenti climatici. Vale la pena di sottolineare che la strategia italiana per il corno d'Africa ci sembra convincente, sostenendo un approccio integrato di diplomazia, cooperazione e negoziato che vada al di là della mera centralità dello strumento militare, ad esempio quella forza ibrida per il Darfur sulla quale sembra ci sia ormai il consenso di tutti. Lo stesso vale per la Somalia, un conflitto ancora difficile, con l'occupazione persistente da parte dell'esercito etiope che però può trovare una svolta, con la recente proposta di Ban Ki-Moon di costituire un contingente di *peacekeepers* ONU, che possa sostenere un processo di pacificazione e mediazione che includa anche le corti islamiche. Abbiamo sentito poco sull'America latina e quasi nulla sul disarmo nucleare, nonostante le sue importanti dichiarazioni fatte in proposito, come anche sulle modalità necessarie per regolamentare il commercio internazionale di armi. Però il tempo è tiranno quindi ci auguriamo di avere in futuro la possibilità di discutere con lei anche di queste questioni, a nostro parere, essenziali per una politica estera coerente, responsabile e solidale. Giacché a fronte di questioni globali, interconnesse, quali la sicurezza, i mutamenti climatici, l'esclusione sociale, il commercio e lo sviluppo sarà a nostro parere necessario superare il concetto e la pratica stessa dell'interesse nazionale, per quella che Peter Singer chiama la prospettiva etica della globalizzazione.

forse non è molto neanche un'ora visto che il nostro Ministro si è dimenticato di dirci che l'Italia ha firmato lo scudo spaziale, che poi veramente è scudo e spada, visto che c'è il primo colpo nucleare; che abbiamo mandato i Carabinieri che fanno parte dell'esercito, in Iraq; del Libano non ha avuto il tempo di dirci nulla, ci ha parlato solo della Siria, dell'Iran e di Hamas, ma non ci ha detto che ci sono gli Stati Uniti e Israele che lavorano con Siniora; non ci ha detto che in Palestina non ci è stato solo l'errore di avere aiutato la formazione dello Stato palestinese, ma anche di avere applicato il boicottaggio allo Stato legittimamente eletto, dopo le elezioni in Palestina, che ha esacerbato i rapporti sociali;

loro considerano le loro basi militari obiettivi di un'eventuale guerra o di attentati terroristici: probabilmente, la vita dei vicentini non gli sta tanto a cuore.

ho apprezzato nella replica anche la definizione che lei ha dato al suo, per altro molto lungo, intervento; fare cioè il punto sulla situazione della politica estera italiana. Mi permetta solo di fare un'osservazione perché il confronto tra lei e l'opposizione sul concetto di politica multilaterale e bilaterale Abbiamo opinioni diverse in materia, non è colpa certamente sua o dell'opposizione, però la preoccupazione che noi abbiamo, quando lei parla di politica multilaterale, è che riteniamo che esistano sedi e luoghi istituzionali in cui il confronto della politica multilaterale porta l'organizzazione stessa a fare una scelta. Avvertiamo, invece, spesso, onorevole Ministro, una politica multilaterale del Governo un po' assembleare e sessantottina, cioè si va in un'istituzione, si fa un dibattito, si espone una linea, ma poi si continua, si ripete in mille occasioni questo dibattito, indebolendo, a nostro giudizio, la stessa concezione di politica multilaterale. L'Afghanistan credo sia un esempio e più ancora Israele e Palestina. Ma questa non è polemica, è solo per capire che non è che rifiutiamo tale linea politica del Governo, ma la riteniamo alla fine quasi un indebolimento, spesso, ci consenta, una fuga dalla realtà per cercare in altre debolezze la non capacità di decisione del Governo italiano. Voglio dire due cose sul Libano e sull'Afghanistan. Lei per la prima volta questa sera, almeno a mia memoria - e confesso che con l'avanzare dell'età anche a me scappa la memoria - ha finalmente detto che UNIFIL l'abbiamo mandata a difesa di Israele; condivido, credo che non sia una posizione condivisa da tutta la maggioranza, ma non è questo il momento di fare polemiche. Se lei voleva, però, fare il punto sulla politica estera italiana, almeno sul Libano, ci consenta, il punto era anche quello di capire in prospettiva del mese di ottobre, che non è lontanissimo, quali iniziative, proposte e atteggiamento intende assumere il Governo italiano sulla materia Libano, atteso che - condividiamo anche in tal caso la posizione del Governo - le forze di interposizione sono lì a mantenere ferma una situazione. Ma la situazione in Libano peggiora, a settembre c'è il problema dell'elezione del Presidente della Repubblica, meglio di me meglio di me lei sa che il problema è che il Libano attende un'iniziativa politica. Per tornare anche in questo caso ad un'altra battuta che raccolgo perché la polemica è un po' il sale del confronto, non è Sarkozy che è diventato l'icona della destra, come lei ha detto, viene da noi accettato quando fa cose che ci piacciono o non viene accettato quando, ad esempio, a La Celle Saint Cloud riunisce tutte le parti. Qui si torna alla polemica precedente del rapporto multilaterale e bilaterale. La Francia intende, all'interno di un sistema multilaterale assumere ogni tanto iniziative assolutamente diverse dal contesto multilaterale, avendo però - se mi consente - la forza politica di imporre o di portare avanti una linea. Fa, cioè, una scelta. Non abbiamo nessun dubbio che anche il Governo italiano in Libano debba fare una sua scelta precisa, anche perché ha questa responsabilità. Per quanto riguarda l'Afghanistan, a ottobre dovremo in Consiglio di sicurezza illustrare o fare una relazione. Mi pare strano che lei non abbia minimamente accennato che il problema nuovo dell'Afghanistan è la debolezza del Pakistan e che la famosa conferenza internazionale che lei spesso ha auspicato è oggi improponibile nella misura in cui manca questo interlocutore pachistano, atteso che ha qualche problema principale al suo interno. Ma venendo alla questione di fondo che riguarda Israele, lei si è presentato, non oggi, ma all'inizio del suo mandato, ribadendo la sua equivicinanza alle forze presenti nel teatro israelo-palestinese. Ovviamente abbiamo replicato legittimamente che, a nostro giudizio, la sicurezza di Israele e la esistenza di Israele sono un problema prioritario. Secondo noi, non vi può essere equivicinanza nell'affermazione di questo principio. È ovvio che, per conseguire questo obiettivo, occorre arrivare ad una trattativa. Ma dov'è il problema da noi sollevato di Hamas? Credo sia in una sua affermazione che ha fatto qui questa sera, che forse l'ha portata a parlare non tanto come Ministro degli esteri, ma come vecchio rappresentante dell'Internazionale socialista: il problema è che Hamas, signor Ministro, è un fenomeno dirompente, ma all'interno del mondo palestinese.

Questo non ha trovato un minimo di condanna da parte del Governo italiano. Non è un problema se Hamas è o può diventare una forza politica, ma è l'accettare una realtà nella quale Hamas ha operato una scelta, ribadendola anche recentemente. Allora oggi non Allora oggi non si può essere né equivicini ad Al Fatah né ad Hamas o fare le affermazioni che lei ha fatto e che hanno creato la forte reazione dell'opposizione. Con questo Hamas non si può, non dico raggiungere un'intesa, ma certamente colloquiare. Lo dico nella convinzione che, prima o poi, con Hamas bisognerà arrivare ad una trattativa. Prima, però, occorre politicamente creare il vuoto attorno ad Hamas

vorrei che lei recepisse dal dibattito dell'Assemblea una forte convergenza da parte di tutte le forze politiche contrarie al piano Ahtisaari, che noi riteniamo ingeneroso e ingiusto nei confronti della Serbia. Lei qui stasera ha dichiarato - e apprezzo questa sua dichiarazione - che l'Italia è amico storico della Serbia. Peccato, devo dire, che nella sua vita politica le sia capitato un momento nel quale è stato molto difficile fare una scelta diversa, bombardando Belgrado. Ma questo fa parte della storia. Se siamo amici della Serbia - e condivido - credo che occorra, innanzitutto, nel dibattito politico cominciare ad affermare un principio per cui i serbi non sono gli unici responsabili della tragedia e dello sfacelo della ex Jugoslavia. Per quanto riguarda il Kosovo, invece, abbiamo due esigenze fondamentali: la prima è quella della sicurezza nazionale. Tutti noi sappiamo e siamo convinti che un Kosovo indipendente sarebbe uno Stato criminale in più, che opera poco lontano dalle coste italiane e, quindi, è un problema fondamentale per noi impedire che nasca uno Stato nelle condizioni in cui si trova oggi il Kosovo. di dover ribadire un inizio di trattativa che aveva visto il Governo italiano assumere una posizione diversa da quella di Ahtisaari. Credo si debba convincere la nazione serba ad accettare il principio del *delinkage*, cioè di cominciare a rompere il legame,

che l'atteggiamento assunto su Israele e Palestina, che resta comunque un momento di fondo, e le molte ambiguità, signor Ministro, che sono anche emerse negli interventi di molti esponenti della maggioranza, dalla senatrice Pisa al senatore Martone, ci convincono che questo Governo sulla politica estera vive momenti di grande difficoltà, che spesso diventano di poca chiarezza. Abbiamo presentato delle proposte di dal Governo) che non erano certamente tese a costruire una contrapposizione tra noi e la maggioranza, ma a cercare di individuare, nel concreto, la possibilità di costruire una grande politica estera di un grande Paese.

che la politica estera del Governo si basa solo su poche parole, poche affermazioni. È meglio non approfondire quello che c'è sotto, perché questo Governo non reggerebbe l'impatto con la realtà.

Forza Italia voterà a favore dei documenti da noi presentati e contro il documento sottoscritto dai Capigruppo della maggioranza, desidero fare alcune riflessioni sulla relazione del Ministro degli affari esteri, che devo francamente giudicare un momento mancato per approfondire le questioni principali, esprimendo quindi un sentimento di rammarico e di delusione. La sua relazione, signor Ministro degli affari non può che essere valutata nei termini di una relazione ordinaria - un elenco delle questioni che il Governo quotidianamente ha nella sua agenda - e soprattutto di una relazione elusiva, cioè concentrata sostanzialmente ad evitare di toccare tasti politicamente dolenti per la sua maggioranza. Avremmo voluto da lei, signor Ministro, nel riprendere il dialogo con il Senato interrotto in un momento forse meno fortunato per il Governo (quando lei, qualche mese fa,

spiegare le sue convinzioni e le sue motivazioni e vide che la sua maggioranza in quell'occasione non condivise la sua relazione e il Governo andò

un elemento che noi abbiamo sottolineato dirimente: un Governo che si presenta alle Camere e che sulla politica estera non ottiene il consenso della propria maggioranza è un Governo che non ha autorevolezza, non ha credibilità ed è un Governo che si deve dimettere. Diamo atto che questo è successo, ma, signor Ministro, non possiamo oggi dare atto che lei ha affrontato nello stesso identico modo tale dibattito. È infatti del tutto evidente

la moratoria della pena di morte, la cooperazione allo sviluppo, il Libano stesso, sono tutte questioni che hanno sempre trovato un largo consenso; ma sulle questioni su cui il consenso non c'è all'interno della sua maggioranza, lei, signor Ministro, si è guardato bene dall'entrare nel merito. Vede, anche lo stesso documento sottoscritto dai Capigruppo della maggioranza è un segnale preciso che la questione era già stata ragionata e decisa prima. È difficile pensare che lei abbia voluto dare la sua relazione anticipata alla maggioranza, poiché il dispositivo con cui la maggioranza approva le sue dichiarazioni è molto semplice: sentite le dichiarazioni del Ministro degli esteri, la maggioranza le approva. Le avevano già sentite queste dichiarazioni, signor Ministro? Il documento è stato depositato prima delle dichiarazioni in quest'Aula e siccome è difficile pensare che la sua maggioranza avesse avuto l'anticipazione, è del tutto legittimo ritenere che lei avesse già

credo chiunque in quest'Aula le riconosca la capacità e l'intelligenza di individuare le questioni della politica più delicate. Quanto alla questione della base

che sul «Corriere della Sera» di ieri c'era un grande articolo che spiegava come alcuni atteggiamenti degli Stati Uniti nei nostri confronti probabilmente andavano imputati a una difficoltà di rapporti. Su tale questione era del tutto chiaro che era necessario da parte sua fare alcune dichiarazioni. Ovviamente non sono state fatte perché avrebbero trovato l'opposizione di una larga parte della sua maggioranza. Come si fa, inoltre, a non ricordare nella sua relazione che ci sono stati 170 parlamentari della sua parte politica che hanno sottoscritto un documento, 170 parlamentari che non hanno avuto alcuna risposta, neanche un accenno, per la paura - questa sì, signor Ministro - di andare anche questa volta ad affrontare un voto difficile del Parlamento? Inoltre, 41 nostri colleghi avevano presentato sull'Afghanistan una posizione che indubbiamente non poteva essere accolta dal Governo. Anche su questo, signor Ministro, lei si è guardato bene dall'intervenire e dal fare riferimenti, evitando che ci possano essere delle lacerazioni. Non è nascondendo la polvere sotto il tappeto, facendo acrobazie o facendo finta che tali problemi non ci siano che si rafforza la credibilità e il prestigio del nostro Paese a livello internazionale. Lei lo sa bene, signor Ministro. Lei e il suo Governo vi trovate oggi di fronte ad un bivio: continuare ad avere un atteggiamento ambiguo, sapendo di non avere una maggioranza in politica estera e di non poter contare sulla credibilità che il nostro Paese dovrebbe avere a livello internazionale, continuare così per mantenere il potere o, viceversa, con uno scatto d'orgoglio cercare di aprire, di allargarsi, di navigare, come lei sa

mozione dei nostri colleghi della maggioranza.

per la sua replica ed anche per il grande equilibrio e l'oggettività di giudizio con cui lei ha espresso il parere del Governo sulle risoluzioni della maggioranza (e questo è naturale), ma anche sulle risoluzioni dell'opposizione. Il ministro D'Alema, iniziando il suo intervento quest'oggi, ha ringraziato il Senato per l'opportunità che gli è stata offerta di informare il Parlamento sull'andamento della nostra politica estera. Voglio aggiungere che negli ultimi dodici mesi l'Aula del Senato ha affrontato, alla presenza del Governo, per ben sei volte temi di politica estera (con dibattiti quasi sempre conclusi con votazioni su numerose mozioni o risoluzioni). Un'informazione puntuale e scrupolosa da parte del Governo al Parlamento in una materia così delicata come la politica estera è doverosa. Ma, altrettanto serenamente, credo vada ricordato che occorrerebbe ancorare sempre questi nostri dibattiti al mutare dell'andamento delle grandi questioni internazionali, all'evoluzione reale degli scenari, alle eventuali modifiche del *modus operandi* degli interventi italiani nelle aree geografiche in cui siamo impegnati. Voglio sottolineare, colleghi senatori, che occorre misura anche nei nostri dibattiti, nel numero delle nostre risoluzioni e delle mozioni che presentiamo al voto dell'Aula del Senato, delle nostre reiterate richieste di ridiscutere, ridiscutere e ridiscutere questioni appena affrontate. Stiamo attenti a non trasformare fruttuose riflessioni sulla politica estera in una serie di schermaglie di politica interna, in un gioco di contrapposizione tra maggioranza e opposizione, in una forma di bipolarismo muscolare ed immaturo. Nel merito, condivido pienamente le dichiarazioni del Ministro degli affari esteri. Penso che il Governo italiano stia sviluppando con saggezza una politica estera autorevole e credibile; una saggezza che si fonda sul basilare principio della coerenza che, come il Senato ben sa, è la prima qualità che si richiede alla politica estera di un grande Paese: coerenza nelle linee strategiche; coerenza nella nostra storica e solida politica di alleanze; coerenza nella presenza nell'ONU; coerenza, infine, con l'aspirazione dei cittadini italiani a vedere il loro Governo impegnato in azioni di pace capaci di consolidare la sicurezza in molte aree del mondo e di portare sicurezza e pace laddove oggi non ci L'Italia deve oggi tener conto di un quadro internazionale instabile e incerto, che non può non condizionare la nostra politica estera e riflettersi anche su tre direttrici cui l'Italia è tradizionalmente ancorata. La prima dalla solidarietà transatlantica, che ci vede alleati liberi, convinti e stabili degli Stati Uniti; ma anche attenti e rispettosi nei confronti dell'ampio dibattito che oggi si sviluppa tra le forze politiche e nell'opinione pubblica di quel Paese e che ha come oggetto la linea e le iniziative della politica estera americana. Signori senatori, ho ascoltato attentamente il dibattito di oggi

ma nessuno ha messo in discussione l'alleanza e il nostro rapporto con gli USA. L'altra direttrice è costituita dal processo d'integrazione europea. Il ministro D'Alema ha ricordato che «la paralisi europea è finita»; voglio aggiungere che la paralisi è finita anche per merito dell'azione del Governo italiano e del suo Ministro degli affari esteri. La terza direttrice - lo ha ben ricordato il senatore Tonini poco fa dalla ricerca di un sempre più elevato livello di stabilizzazione e di pace nel Mediterraneo. Il Mediterraneo rappresenta una straordinaria opportunità storica per il nostro Paese; un mare interno che collega l'Europa al Nord Africa e al Medio Oriente, un'area che per molti secoli ha vissuto una condizione di forte marginalità e che negli ultimi tempi sta diventando un luogo di straordinaria importanza per scambi commerciali, traffici economici, collaborazione culturale e politica. Per l'Italia, e in primo luogo per il nostro Mezzogiorno, il Mediterraneo può essere una grandissima occasione; ma perché lo sia veramente occorre che a tutti i Paesi che vi si affacciano sia garantita stabilità e convivenza pacifica. L'Italia sente come una sua missione la pace e la stabilità del Mediterraneo. Questa è la radice della sua continua e attenta iniziativa politica, ma anche della nostra presenza militare di pace in un'area delicata come quella del Libano e, più a distanza, dell'Afghanistan. Sono scelte di politica estera che hanno fatto crescere l'autorevolezza e la credibilità del nostro Paese e hanno portato l'Italia ad essere eletta, con grande consenso, nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il compito dell'Italia è di rafforzare il multilateralismo, non certo di indebolirlo. Ma per poter dispiegare con efficacia l'azione del nostro Paese, occorre assumersi responsabilità corrispondenti: ed è quello che l'Italia ha fatto, sta facendo e farà nelle rilevanti missioni internazionali cui partecipa. C'è uno stretto legame tra l'assunzione di responsabilità, anche militari, e la pace. Anzi, sono proprio le missioni di pace ad essere l'unico impegno militare che il nostro Paese può assumere, se vuole essere fedele all'articolo 11 della Costituzione. Questa cornice è per noi inviolabile. Ma sappiamo bene che la pace, contro coloro che fomentano terrore e violenze, si difende anche con l'uso legittimo della forza. Lo ha ricordato poco tempo fa il ministro della difesa, Parisi: quello italiano - ha detto il ministro Parisi - non è un "Governo pacifista, se pacifismo significa il rifiuto pregiudiziale dell'uso della forza legittima contro la violenza ingiusta". Io aggiungo che quello italiano è un Governo che opera per la pace e lo fa anche con le missioni internazionali dei suoi soldati, che oggi io voglio qui ringraziare in Aula per il loro sacrificio, per il loro impegno, per la straordinaria competenza professionale e per l'umanità con la quale svolgono la loro missione. Concludo rivolgendomi all'opposizione, cui vorrei ricordare che oggi nel nostro Paese c'è una condivisione molto larga sulle grandi direttrici della politica estera italiana: condivisione sulla volontà di pace e di stabilità internazionale; sulla necessità di una forte solidarietà transatlantica; sulla lotta al terrorismo internazionale; sul forte impulso da imprimere al processo di integrazione europea; sulla necessità di una decisa iniziativa politica per la stabilizzazione e per la pace nel Mediterraneo. Tutti sappiamo che queste tre grandi stelle polari della nostra politica estera sono oggi quanto mai attuali, ma anche caratterizzate da elementi incertezza. E, attorno ad esse, si è sviluppato un forte dibattito. Ma è un dibattito sul "come", non sul "se". Il mio Il mio invito all'opposizione è a tenere conto di questo quadro generale e a non attribuire al Governo italiano la responsabilità delle incertezze e delle debolezze dello scenario internazionale. È possibile che su singoli punti della politica estera del Governo sussistano dissensi; ma il mio invito è che non vengano utilizzati dissensi su singole questioni per rimettere in discussione i principali fondamenti della politica estera del nostro Paese. Il Gruppo dell'Ulivo voterà a favore della risoluzione della maggioranza e vuole adesso formulare auguri di buon lavoro a lei, ministro D'Alema, e a tutto il Governo.

riferendosi agli impegni assunti dall'Italia nelle missioni internazionali i supporti logistici sono quelli delle Forze armate italiane e noi siamo a favore della logistica delle Forze armate italiane. Per quanto riguarda la proposta La caserma "Ederle" è una caserma italiana a tutti gli effetti e quindi si intende che supporti e confermi anche quel tipo di accordo.

D'Alema, che «esprime un parere contrario; tanto più che la parte positiva di questa proposta di risoluzione, cioè ribadire il valore del rapporto con gli Stati Uniti mi pare assorbito dal parere favorevole sulla precedente proposta di risoluzione che va in questo senso». Il dispositivo della mia risoluzione recita: «esprime apprezzamento nei confronti delle posizioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Governo in occasione degli incontri e dei colloqui avuti con il Presidente degli Stati Uniti e con il Primo Ministro di Israele», mentre nella precedente

del ruolo svolto dall'Italia, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, nel processo di pace con particolare riferimento alla questione medio-orientale». Ora, non è che voglia che il Governo torni sui suoi pensieri,

Per quanto riguarda quest'ultima sua riflessione, credo che non ce l'abbia nessuno. Comunque, la proposta di risoluzione ha avuto il parere contrario del Governo.

per l'atteggiamento dei Capi di Stato nei confronti del nostro ruolo nelle missioni internazionali e altro è esprimere censura nei confronti di chi ha detto che il Presidente degli Stati Uniti ha le mani sporche di sangue.

parere contrario del Governo.

vi è l'appello di 41 senatori che richiedono una linea di discontinuità rispetto all'Afghanistan e nel dispositivo si apprezza la linea tenuta dal Governo in Afghanistan.

La proposta finora fatta dal senatore Boccia era: due voti. Il primo per tutta la premessa;

una dichiarazione di stampa, che ho sottoscritto e ribadisco in questa sede. Non capisco, però, quale valore normativo possa avere approvare o meno la notizia che è stata presentata una dichiarazione alla stampa. Ben diversa è la proposta, che condivido, del senatore Boccia e che corrisponde al parere del Governo, di separare l'apprezzamento per la politica estera del Governo dalla premessa. Oltretutto, vorrei ricordare che il Parlamento ha deciso che sulle missioni in Afghanistan si voterà in altra occasione e quella è la sede in cui ciascuno di noi, ascoltato il Governo, farà valere il suo giudizio. Onestamente, non capisco come si possa votare su una dichiarazione alla stampa; che cosa si vota? La veridicità? Sì, è vero; l'abbiamo fatta.

che ha deciso dell'ammissibilità o meno e noi ne prendiamo atto. A questo punto, però, come già diceva il senatore Sodano poco fa, noi chiediamo per ovvi motivi, peraltro conseguenti alla sua valutazione di ammissibilità, non due, ma tre votazioni; e spiego

che spero superato e che comunque mi ha in qualche modo...

svolto un alto dibattito di politica estera, sia come maggioranza sia come opposizione, su una relazione di grande spessore del Governo, stiamo votando una premessa che si basa sulla notizia giornalistica di un appello rivolto da 41 senatori.

Presidente, sono disposto ad accettare una certa forzatura della logica umana, connessa ai lavori di un'Aula parlamentare; però, se sarò costretto ad esprimermi su un anacoluto

Signor Presidente, onorevoli colleghi, premesso che giustamente la Presidenza ha ha sollecitato l'Aula e ciascuno di noi al rispetto del Regolamento che attribuisce al Presidente la decisione ultima circa le modalità di votazioni delle risoluzioni, la mia opinione è la seguente e la sottopongo all'attenzione dell'Aula: abbiamo svolto sulla politica estera, nel corso di questo pomeriggio, una discussione assai importante

Il Governo ha certamente fatto cosa utile mostrando attenzione per ognuna delle proposte

Accade, tuttavia, che, per ragioni che posso comprendere e che non contesto nel merito, che venga presentata una proposta che non isola nel documento la parte su cui il Governo ha espresso parere favorevole da tutto il resto (su

La Presidenza la considera ammissibile: non contesto la Presidenza, anche se è del tutto evidente che nella seconda votazione si mette ai voti un anacoluto. È chiaro che,

voterà contro la prima parte, non tanto e non solo per il contenuto, ma per il non senso di mettere in votazione una dichiarazione di alcuni colleghi alla stampa.

*corpus* del testo. Quindi, sono tre le proposte. Gradirei che lei ci dicesse chiaramente su cosa dobbiamo votare. Quanto poi al fatto che alcune votazioni siano assurde o meno, questo lo lascerei al buonsenso dei colleghi, perché non mi pare giusto anticipare alcuni giudizi di questa natura, atteso che non è la prima volta che si votano per parti

Morando. Rileggendo quello che ha dichiarato il Governo, per la proposta di risoluzione n. 11 esprime parere favorevole sul dispositivo, che mi pare una sintesi felice, dove si legge: «approva la politica estera seguita dal Governo nella missione in Afghanistan». Mi sembra che regga perfettamente in forma isolata e che ci sia, conformemente, un parere favorevole sul dispositivo.

parere contrario del Governo.

Che valore hanno le risoluzioni del Senato, signor Presidente, lei che ci deve tutelare? Vale qualcosa il voto di prima o è stata una cosa fatta così, giusto tra amici? Vale qualcosa, secondo lei, che è il Presidente del Senato, che è il garante della forza del voto che avviene in quest'Aula, il fatto che quest'Aula abbia bocciato l'approvazione della politica estera del Governo o non vale nulla? Credo sia una domanda che dobbiamo assolutamente porci, a cui lei deve dare una risposta in questo momento, altrimenti vuol dire che stiamo qui a prendere in giro non soltanto noi stessi, ma soprattutto il popolo italiano. E' stata respinta una risoluzione. Prima di andare avanti, signor Presidente, le chiedo che valore ha questa risoluzione.

la prima riguarda sicuramente il merito; è evidente che, avendo l'Assemblea approvato la prima proposta di risoluzione, nella quale si approva la linea di politica estera del Governo, non poteva

Sicuramente vi è stato un errore, per cui le chiederei la cortesia, con calma, prima di certificare il risultato, poiché è possibile fare una verifica visiva dei tabelloni, di verificare se al risultato conclamato dalla comunicazione corrisponde effettivamente il risultato del voto. Noi pensiamo che vi sia un errore materiale, a parte questo, vorrei che fosse chiaro ai colleghi che schiamazzano che il primo voto ha approvato la linea di politica estera del Governo. Quindi, il secondo voto non ha alcuna importanza!

io credo che la seduta, nella sua "stravaganza", abbia registrato due votazioni componibili. Il fatto che sulla politica estera del Governo si sia registrata la maggioranza del Senato è ineccepibile. Come tutti sappiamo, però, la politica estera del Governo si sostanzia in alcuni fatti di particolare rilievo, alcuni dei quali hanno creato e creano problemi all'interno della maggioranza di Governo: uno è stato giocato

Questa maggioranza ha bocciato la politica del Governo in Afghanistan. Cosa c'è di sconvolgente, collega Boccia? È stata bocciata una parte della politica estera. Niente di strano, ma questo fatto nelle cancellerie internazionali è rilevante, altro che storie! *(Applausi dai Gruppi UDC e FI).* Nel resto del mondo conta moltissimo. Da domani la gente vorrà sapere cosa è successo e possiamo dire che c'è stato un equivoco? Che alcuni colleghi non hanno capito cosa facevano?

Grazie, signor Presidente, molto gentile per avermi dato la parola, anche se un po' in ritardo. Vorrei prima di tutto darle atto della correttezza dei suoi comportamenti. Il voto è ineccepibile. Vorrei ripetere che quest'Aula ha chiaramente approvato la politica estera del Governo in generale, ma ha espresso voto contrario sulla politica estera del nostro Governo in Afghanistan. Credo che la cosa non sia politicamente irrilevante. Credo che il Governo abbia bisogno di riflettere per capire se accetta un voto favorevole sulla sua politica estera, ma non sulla politica estera in Afghanistan o se la bocciatura della sua politica estera in Afghanistan lo induce a considerare come politicamente troppo fragile e insostenibile l'approvazione data in generale di una visione ampia ma confusa, ampia ma generica, ampia ma astratta, della sua politica. Quindi, mi domando se non sarebbe più utile, a questo punto, sospendere la seduta e invitare il Governo a fare le sue riflessioni sul significato politico di questo voto, per comunicarci poi quali conseguenze intende trarne. punto all'ordine del giorno e continuare con le votazioni mi sembra violare quanto chiaramente è avvenuto in quest'Aula. Un pezzo fondamentale della politica estera di questo Governo è stato bocciato. Non è come se non fosse successo nulla. È accaduto un fatto politicamente significativo. Il Governo deve riflettere su questo fatto. Credo che sia improponibile continuare con i lavori.

dopo un voto del quale ovviamente non possiamo contestare l'oggettività, sul fatto che poc'anzi, all'unanimità, o quasi unanimità, ma sarà facile rintracciare i tabulati (era di certo quasi tutto verde il pannello il Senato ha approvato la proposta di risoluzione n. 5 dei senatori Mantica, Pianetta e Antonione, il cui dispositivo, lo ricordo a tutti, recita: «Il Senato, impegna il Governo: a confermare l'impegno e la presenza in Afghanistan, pur profilandosi lunga e complessa, per la costruzione della pace e della stabilità». Ora, se i nostri precedenti e quindi le decisioni che sono state adottate all'inizio dal presidente Marini, e che ovviamente non contestiamo, fossero stati tali da poter stabilire un regime di preclusione, è ovvio che l'unanimità del Senato, che conferma l'impegno e la presenza in Afghanistan, pur profilandosi lunga e complessa per la costruzione della pace e della stabilità, è un giudizio nettamente positivo sull'azione del Governo ed anzi un incoraggiamento, pur nella lunghezza e complessità della costruzione, a perdurare in questo compito. Credo quindi che non dobbiamo occuparci del fatto che sia stato successivamente espresso un voto, che non contesto nella sua oggettività ma che certamente è quello che è, ma dovremmo piuttosto preoccuparci del fatto che il voto susseguente ha smentito un altro assunto all'unanimità del Senato, che è nettamente in contrasto con il secondo. Signor Presidente, non metto in discussione la legittimità del voto, ma

del percorso logico‑procedurale che abbiamo seguito per la votazione della proposta di risoluzione n. 11. L'Aula si è avvitata per 15-20 minuti sulle modalità del voto di questa proposta di risoluzione: se per parti separate, se per intero, se per due o tre parti. Molti esponenti della maggioranza si sono pronunziati su come volevano che si votasse questa risoluzione, di nessuno, signor Presidente, si è espresso un giudizio di presunta inammissibilità della stessa.

quindi di non arrampicarvi sugli specchi e prendete atto che il Senato, con il voto di poco fa, ha bocciato la politica estera del Governo in Afghanistan e il Ministro degli esteri ne prenda atto.

alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa» le parole «con particolare riferimento alle sue radici giudaico-cristiane». Il Ministro, nell'esprimere il suo parere contrario, ha affermato: «(...) perché il Governo intende partecipare alla conferenza intergovernativa sulla base del mandato approvato dal Consiglio europeo, che non prevede una correzione del preambolo».

14 dicembre 2006, avente ad oggetto un grosso problema che insiste sull'aeroporto bergamasco di Orio al Serio, dove non sono state probabilmente rispettate alcune regole imposte dall'ENAV, soprattutto, non è stato rispettato un accordo programmatico concordato dal Governo nel territorio e con la Regione Lombardia. Dal momento che si stanno rivolgendo a me diversi sindaci del territorio in cui rilevano queste gravi

in cui hanno perso la vita alcuni cittadini pugliesi: il bilancio delle ultime ore, purtroppo, vede 373 ustionati e 3700 sfollati. Nell'interrogazione i senatori chiedono che il Governo venga a riferire al più presto in quest'Aula.